L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signor Presidente, ho chiesto la parola innanzi tutto per annunciare che i senatori del Partito Democratico presenteranno oggi stesso un atto formale di solidarietà al ministro Cécile Kyenge Presidente, noi consideriamo molto gravi le espressioni che il senatore Roberto Calderoli, che mi dispiace non vedere adesso in Aula che è Vice Presidente del Senato, riteniamo che lo stesso senatore abbia sbagliato a definire quelle parole in un'intervista una "battuta infelice",

quando sta in Senato e non esserlo più in tutte le altre sedi nelle quali parla e fa politica. Quando un Vice Presidente del Senato insulta gravemente un Ministro della Repubblica sussistono evidenti ragioni

in virtù del Regolamento del Senato, la vice presidente Rosi Mauro rimase al suo posto, nonostante la richiesta di dimissioni le fosse stata rivolta da gran parte dei Gruppi ed anche dal suo stesso partito. Il senatore Calderoli deve riflettere su quanto la mancanza di una previsione regolamentare e di una sanzione di sfiducia nei confronti dei Vice Presidenti li carichi di maggiori responsabilità e li obblighi a tenere comportamenti consoni alla loro carica. La frase di Roberto Calderoli nei confronti della ministro Kyenge non può essere considerata una polemica politica: non contiene una valutazione istituzionale e neanche un giudizio di merito nei confronti dell'azione di un Ministro, la cui politica sullo *ius soli* noi condividiamo pienamente e chiediamo diventi al più presto legge dello Stato. Quella frase è solo un insulto razzista, la cui volgarità è molto più grave perché rivolta contro una donna. in nessun altro Paese d'Europa un Vice Presidente del Senato potrebbe usare espressioni simili rivolgendosi a un Ministro del suo Paese, o a un cittadino, senza essere sanzionato, in alcuni Paesi, anche penalmente. Signori senatori, questi episodi alimentano il distacco crescente nei confronti della politica. Né si stupisca la Lega Nord per la perdita progressiva di consensi elettorali. Gli italiani non ne possono più di insulti, urla, volgarità, trabocchetti e manovre destabilizzanti. Pochi giorni fa, io stesso in quest'Aula ho apprezzato il senatore Calderoli per la capacità con la quale aveva esercitato il suo turno di Presidenza. E lo ricordo per sottolineare l'assenza di qualsiasi pregiudizio negativo politico nei suoi confronti. La forte censura dei senatori del Partito Democratico per l'ingiuria con cui si è rivolto al ministro Kyenge non ha quindi alcuna origine politica di parte, ma noi vogliamo, signor Presidente, che la politica sappia ritrovare credibilità, e sappia farlo comportandosi con onore. Per questi motivi chiediamo al senatore Calderoli di dimostrare di possedere, oltre all'abilità di Aula, anche il necessario senso delle istituzioni, e gli chiediamo di rassegnare le dimissioni da Vice Presidente. *(Applausi Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono i luoghi della democrazia, ma il prestigio del Senato non sta nella bellezza delle mura di Palazzo Madama e dei velluti su cui noi sediamo in quest'Aula: il prestigio del Senato lo determiniamo noi senatori, con il nostro comportamento dentro e fuori dell'Aula. Ciascuno di noi, a partire da chi ricopre la carica di Vice Presidente del Senato, deve sentire su se stesso la responsabilità della difesa dell'istituzione di cui è *pro tempore* componente. Grazie, signor

vorrei esprimere, a nome mio e di tutte le senatrici e i senatori del Gruppo Misto, la piena solidarietà alla ministra Kyenge.

Questa è una ferita molto forte per il nostro Paese e per la credibilità delle istituzioni. Per questo, noi chiediamo a gran voce

offesa razzista, l'esempio più classico del pregiudizio razziale. Questo in un Paese, torno a ripeterlo, in cui con allarme segnaliamo ogni giorno una ripresa di campagne

l'offesa del senatore Calderoli è su tutte le pagine dei giornali esteri, e questo è un grave danno all'immagine del nostro Paese.

delle istituzioni. Non vorrei che queste offese siano state utilizzate per alimentare facili consensi

poter formalizzare mozioni di sfiducia, perché siamo in un'ipotesi di Regolamento completamente diversa, però quest'Assemblea non può che - spero unanimemente - chiedere al senatore Calderoli,

non possiamo sottacere è che volutamente non si voglia riconoscere il suo essere pienamente cittadina italiana e quindi il suo pieno diritto di essere nominata Ministro nel Governo del nostro Paese.

ferma solidarietà al ministro Cécile Kyenge per le parole di inusitata gravità che sono state pronunciate dal Vice Presidente di quest'Aula, senatore Calderoli, nei giorni scorsi. Parole che rappresentano veri e propri insulti razzisti, che - non dimentichiamolo - sono reato a norma di una legge approvata da questa stessa Aula nel 2003. Parole che sono pesanti e che creano grave disagio in tutti noi rappresentanti del popolo italiano.

le sue affermazioni, né ha senso far finta di cospargersi il capo per correggere affermazioni che da nessuna parte d'Europa sarebbero accettate. l'Italia, di fronte a parole che offendono le istituzioni e contrastano gravemente con l'affermazione dei diritti inalienabili di ogni persona, chiede al senatore Calderoli di dimettersi immediatamente dall'alto incarico di Vice Presidente del Senato della Repubblica. Inoltre, signor Presidente, mi rivolgo a lei: il Gruppo di Scelta Civica, qualora il senatore Calderoli non provvedesse a tale necessario atto, di assumere ogni deliberazione affinché egli non presieda più quest'Assemblea e, soprattutto, non vengano più affidati incarichi che vedano la rappresentanza ufficiale del Senato della Repubblica ad una persona che ha fatto affermazioni che contrastano gravemente con i principi costituzionali. Scelta Civica ritiene che sia importante andare in questo momento a ribadire queste cose con la forza necessaria, perché il nostro Paese ha bisogno di sentirsi unito intorno a valori fondanti e la questione che oggi è in gioco è elemento fondante e decisivo.

abbiamo insistito sulla necessità di fare un salto di qualità perché qualunque espressione infelicissima e sgradevolissima che richiami l'offesa del razzismo nasce da ignoranza, leggerezza e trascuratezza nei confronti dei valori e della dignità delle persone. Per noi questo è cultura. È cultura, per esempio, l'atteggiamento che ha tenuto il Ministro in questione, che, per quello so e per quello che abbiamo letto, ha dimostrato grande signorilità nel rispondere al collega Calderoli

Noi rimarchiamo che vi è in Italia, per responsabilità vostra (dico vostra), un'assenza vera su questioni che sono drammatiche, perché può essere oggi razzismo, può essere domani femminicidio, può essere dopodomani omofobia, ma tutto questo nasce da assenza di cultura. E noi, negli ultimi decenni, piuttosto che investire in cultura su tutti i fronti e con qualunque maggioranza, abbiamo tolto soldi all'istruzione pubblica, alla cultura, alle politiche di integrazione: con qualunque maggioranza

vorremmo andare oltre: vorremmo che questo Parlamento si facesse carico ora di parole sgradevoli, ora di gesti assolutamente offensivi rivolti al pubblico (e mi ricordo che un altro Presidente del Senato è stato immortalato con uno scatto fotografico mentre faceva capire che cosa pensava della gente che lo denigrava), soprattutto che tutti quanti riconquistassimo un tenore di civiltà. Ebbene, tutto questo lo possiamo fare soltanto se, al di là dell'ipocrisia del momento, andiamo oltre la richiesta di semplici, circostanziate e contingenti dimissioni, perché l'Italia è capace di far altro, sempre che noi qua dentro ci si impegni a farlo. E allora investiamo in cultura, investiamo in pubblica istruzione! *(Applausi dite invece che in Commissione pubblica istruzione non si trovano pochi milioni per affrontare la questione degli inidonei nella scuola. Certo, il Ministro ha dimostrato grande signorilità, e tutta questa signorilità è espressione di cultura e di moralità. Ma questo è possibile quando non sei alla disperazione, quando non sei nella miseria, e per nostra fortuna il Ministro ha fatto capire che è di altra pasta. Vorremmo che tutti gli italiani fossero messi in condizione di poter pensare a queste parole, che appartengono ad ognuno di noi, come a qualcosa del passato e non di un presente che ritorna!

questo dibattito fa male alle istituzioni e alla civiltà delle istituzioni. Fa male perché nel 2013 dubito che vi siano Parlamenti in Europa che si occupino dell'attacco di un Vice Presidente del Senato a un Ministro o comunque ad un cittadino della medesima Repubblica con le parole che sono state usate. Non basta in questo caso manifestare una solidarietà pelosa e passiva: serve qualcosa di più, come è già stato ricordato, a cominciare dal collega presidente Zanda. Fa male alla civiltà giuridica delle istituzioni perché, nel caso in cui un'alta carica dello Stato si fosse trovata in questa condizione, avrebbe evitato ad una istituzione di discuterne, muovendosi prima che fosse richiamato dentro all'istituzione che presiede peraltro ottimamente e più volte - a rendere ragione di un comportamento. Quest'Assemblea, signor Presidente, ha discusso recentemente e in passato di tutto: recentemente, è stato ricordato dal presidente Morra, della Convenzione di Istanbul; abbiamo ratificato tutte le varie e diverse tipologie di trattati inneggianti ai diritti umani e ai diritti civili. Non ci manca che l'assunzione o la ratifica del galateo di Giovanni Della Casa, del quale comunque conviene la lettura. Il punto è che, se il senatore Calderoli non si riconosce nella diversità e alla diversità non riconosce uguaglianza di diritti, noi azzeriamo secoli di lotta per la libertà. Questo è il punto, tanto più grave se proviene dal Vice Presidente del Senato. In quest'Aula alcuni anni fa risuonarono le parole di un senatore della Repubblica, Mario Luzi, che, prima di andarsene (su questi scranni rimase pochissimo, essendo già molto anziano quando venne nominato dal presidente della Repubblica Ciampi), lasciò poche parole, più o meno le seguenti: la libertà è una palestra nella quale conviene andare ogni giorno, perché chi non frequenta quella palestra rischia di inaridirsi. Quest'Aula non può chiedere in maniera formale le dimissioni del Vice Presidente del Senato, perché

una richiesta corale dell'intero Parlamento che vada in questa direzione, perché oggi parliamo di condivisione o no di un diritto comune e di valori condivisi. Quindi, non può esserci soltanto una parte del Senato

anche il nostro Gruppo esprime incondizionata solidarietà e, se ci è consentito, anche amicizia alla ministra Cécile Kyenge, bersaglio di qualcosa di più di parole infelici: bersaglio di una sguaiata esplosione di razzismo, ha detto chi mi ha preceduto. Forse, nella speranza che il linguaggio di comizio non faccia testo fuori da quel contesto, un collega un collega - se me lo consentite, un amico - che da molti anni avevo sempre stimato si è abbandonato ad un linguaggio inammissibile nei confronti di qualsiasi signora. Definire la ministra Cécile Kyenge "un orango" è un'espressione che squalifica qualunque argomento possa essere stato portato contro la politica di di tale rappresentante del Governo. Non più tardi di un mese, un mese e mezzo fa, la politica del Ministro, le sue dichiarazioni programmatiche in merito a intenzioni legislative erano state oggetto sul «Corriere della Sera» di un editoriale di Giovanni Sartori

(odiosa perché istiga all'odio). Allora, da questo punto di vista mi sarei

con lo spirito e l'improntitudine che talvolta lo caratterizza e per la quale molti di noi lo hanno apprezzato: non ero io, era uno che mi somiglia; ho già mandato a nome di tutto il Senato

Speriamo che i colleghi della Lega riescano ad ottenere da Calderoli un modo garbato perché il Senato non sia più prigioniero di una vicenda che è sgradevole, non già per il Senato ma per il nostro Paese e per la nostra generazione,

a me sembra che si sia trovata un po' una scusa con la vicenda infelicissima dell'amico Calderoli.

credo che tutti o tanti di quelli che hanno parlato dovrebbero ricordarsi qual è il linguaggio che oggi si usa nei confronti dell'avversario politico.

ovvero aggredire la collega Carfagna. Io non ho sentito nessuna voce, non ho sentito nessuno che si sia lamentato.

la rimozione dall'incarico a cui quella persona è destinata. Stenderei quindi un velo pietoso su questo. Mi dolgo e mi dispiace per la Ministra, non meritava questo, anche perché sta lavorando bene, ancorché su progetti che noi non condividiamo, ma che saranno oggetto di discussione in quest'Aula. Mi dispiace per il vicepresidente Calderoli, ma insisto e ripeto che è un fatto che deve rimanere fuori da quest'Aula. Il Vice Presidente oggi è assente, e mi dispiace che non assista a questo

ma non sarà il primo né l'ultimo. Ritengo invece - e qui riprendo una parola del collega Zanda - che la politica dovrebbe continuare a dimostrare credibilità: con questi dibattiti non credo che lo stiamo facendo.

Presidente, potrei esordire con una frase abbastanza nota: sento che in quest'Aula tutto ci è ostile tranne la vostra personale cortesia. fare un ragionamento pacato, definendo alcune questioni. L'assenza del vice presidente Calderoli era stata già comunicata: c'è una segreteria politica in atto a Milano, quindi non è strumentale, ma precedente a quello di cui oggi si sta discutendo. I colleghi che sono intervenuti hanno evidenziato un fatto

Tutti noi sappiamo cosa sia la stampa estera e cosa siano i corrispondenti esteri: il corrispondente estero a Roma o scrive qualcosa di interessante o viene richiamato. E quando noi forniamo materiale

Il corrispondente prende i nostri bei giornali, possibilmente scandalistici, copia e incolla, taglia e cuce e fa il suo articolo. Inutile poi dire che anche dall'estero veniamo trattati come veniamo trattati. Se poi facciamo anche confusione, volontaria o involontaria, attribuendo dei fatti (come ha fatto il collega Morra)

mancanza di indipendenza. Gli apprezzamenti sono stati fatti, mi sembra, anche in questa sede. L'altro livello è quello politico‑partitico. Ognuno di noi, ognuno di voi, si trova in momenti particolari: si fanno campagne elettorali dove i colpi bassi girano spesso e volentieri,

Ma, ripeto, siamo in due ambiti completamente diversi. In questa seconda veste, se vogliamo, possiamo ammettere anche noi che il collega Calderoli ha probabilmente ecceduto,

scuse. Mescolare l'aspetto istituzionale con quello partitico-politico sarebbe un grave errore. Non è il caso di scomodare Voltaire in quest'Aula, ma richiamare il principio dei due frasi offensive in questi ultimi periodi ne abbiamo sentite in misura debordante. Non credo che Grillo possa insegnare niente a nessuno in fatto di stile o di *bon ton*,

non abbiamo mai sentito sollevarsi un'indignazione come quella che stiamo ascoltando in questi giorni e oggi in quest'Aula. Colleghi, due pesi e due misure. Devo dirlo, anche se è qualcosa che ci tocca e ci fa male, ma una persona della Lega probabilmente sarà bollata a vita per un epiteto giocato. E stampa e ristampa, a cascata, utilizzando un brutto appellativo, probabilmente Renzo Bossi, unico consigliere regionale d'Italia dimessosi senza aver ricevuto nemmeno un avviso di garanzia, ma per quanto è successo attorno a se stesso, l'appellativo "trota" non se lo non se lo toglierà più per tutta la vita. *(Commenti).* Non abbiamo sentito - scusate, colleghi - una persona richiamare anche in questo caso la dignità del soggetto che è stato preso in mezzo. Per noi, per quanto concerne il Gruppo della Lega, il caso è chiuso. Siamo convinti che c'è stata un'intemperanza; ci sono state delle pubbliche scuse. Inviterei però tutti i colleghi

chi in buona fede, chi ingenuamente vi sia caduto - serva per coprire qualcosa che sta accadendo sotto i nostri occhi, ma da cui forse è meglio deviare l'attenzione. Ed è una brutta vicenda di rapporti internazionali tra l'Italia e il Kazakistan.

non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: per la Regione Friuli-Venezia Giulia: Lorenzo Battista, Bernabò Bocca, Isabella De Monte, Alessandro Maran, Carlo Pegorer, Francesco Russo e Lodovico Sonego. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Vorrei qui ricordare che il progetto per la realizzazione di questo velivolo è frutto di un accordo tra gli Stati Uniti e otto Paesi *partner*, tra cui l'Italia, che prevede la realizzazione di 3.173 velivoli, per un costo complessivo stimato di 396 miliardi di dollari, anche se - questo è uno dei primi elementi critici - nessuno, allo stato attuale, è in grado di quantificare il costo finale dell'intero progetto. Ogni singolo aereo oggi è stimato comunque intorno ai 190 milioni di dollari.

stanno in qualche modo mettendo in discussione la partecipazione a questo programma. La Gran Bretagna deciderà il numero degli aerei acquistati solo dopo la pubblicazione del *Defence and security review*, nel 2015. L'Olanda ha avviato un'inchiesta parlamentare. L'Australia non userà gli F-35 come piattaforma esclusiva. La Turchia ha rinviato l'acquisto dei primi F-35. La Norvegia, dove vi è un dibattito molto acceso, acceso, varie volte ha ventilato l'ipotesi di ripensare le sue scelte sugli F-35. La Danimarca ha riaperto la gara, per decidere entro il 2015 di quale aereo dotarsi.

Governo: uno studio indipendente (Kpgm) ed altri organi di controllo pubblici hanno infatti stabilito che il costo complessivo in 40 anni, includendo anche l'uso e la manutenzione, è di oltre 45 miliardi di dollari,

Queste sono le cifre di cui oggi stiamo parlando.

di *peacekeeping* per le forze armate;

Grazie

Signor Presidente del Senato, signori senatori, signori del Governo, fin dal termine della passata legislatura la vicenda dei cacciabombardieri d'assalto F-35 era venuta all'attenzione del Parlamento e, inesorabile, si è ripresentata all'inizio di questa legislatura come uno dei temi più emblematici e contrastati. Il 6 giugno di quest'anno è stata pubblicata, e unita agli atti della seduta del Senato, prima ancora che se ne parlasse in Aula alla Camera dei deputati, con la firma di oltre 20 senatori, la mozione sugli F-35 in discussione oggi e a mia prima firma. L'intera vicenda, delicata e controversa anche per gli equilibri tra i Gruppi parlamentari, può essere affrontata e discussa almeno sotto tre aspetti. Il primo livello, per certi versi più chiaro e netto, è quello del richiamo alla pace, al pacifismo, alla costruzione della pace. talmente chiaro e netto da potersi ritenere preclusivo di ogni altra considerazione nei confronti di uno strumento bellico, come oggettivamente è un cacciabombardiere d'assalto. Ma non mi voglio dilungare sul punto, peraltro lampante, ritenendo invece di dover affrontare in questa sede gli altri aspetti più dibattuti della questione, proprio per illustrare il motivo per cui il programma degli F-35 dovrebbe essere sospeso immediatamente. - pesanti critiche - al progetto degli F-35 provengono dallo stesso mondo militare-industriale. Sono ben note, direi ormai notorie, le peripezie (anche gravi) che stanno accompagnando la nascita di questo progetto, tanto da aver determinato il ripensamento, il ridimensionamento o addirittura l'annullamento della propria partecipazione al programma da parte della maggioranza degli Stati partecipanti, a seguito soprattutto dei costi esorbitanti e in continua inarrestabile ascesa, per di più in presenza di criticità tecnologiche e tecniche preoccupanti e di assoluto rilievo, che hanno condotto persino il Pentagono e lo statunitense GAO (*Government accountability office*) a far segnare il passo. Ma è soprattutto dall'interno del mondo militare italiano che giungono serrate e convinte critiche. Il capo di Stato maggiore delle Forze NATO del Sud-Europa, già comandante della missione NATO-KFOR nel 2002-2003, il generale Fabio Mini, ha pubblicamente denunziato il velleitarismo del programma, auspicando invece un modello nuovo e diverso di difesa, integrato come minimo a livello europeo, che in questa prospettiva, pur salvaguardando qualità e quantità, potrebbe condurre almeno ad un dimezzamento dell'attuale bilancio della Difesa italiana. E sempre restando al cacciabombardiere d'assalto F-35, mi limito a ricordare quanto ulteriormente denunciato dalla cosiddetta Bibbia dell'Aeronautica, "Aviation Week", che ha parlato di notevoli inadeguatezze tecniche, tanto che si è pure scritto di un caccia costoso, problematico e inaffidabile. Ma senza volermi addentrare in più specialistiche disquisizioni e valutazioni tecniche, registro l'esistenza di alternative ritenute più affidabili, meno costose e con maggiori ricadute sia tecnologiche che economiche, come il programma Eurofighter o la scelta prioritaria di puntare su una certa tipologia di elicotteri, opzioni sulle quali non svolgo alcuna considerazione. Questa ultima riflessione mi consente di passare al terzo livello della vicenda, quello attinente ai presunti vantaggi economici e occupazionali che sarebbero garantiti dal programma F-35. Ora, a parte il fatto che i dati forniti dalle aziende interessate risalgono ad oltre un lustro fa (un periodo eccessivamente ampio rispetto alle vicende finanziarie e alle sventure tecniche dei prototipi degli ultimi anni), una risposta negativa viene imposta da una duplice elementare considerazione. In primo luogo, i costi del programma, nella loro enormità, sono in continua e imprevedibile ascesa, aggravata dal fatto che già si è verificato a livello internazionale un occultamento dei dati finanziari, particolarmente in riferimento all'uso e alla manutenzione degli aerei. luogo, in questo momento di crisi economica, occupazionale, finanziaria che ha colpito anche l'Italia e in un momento storico in cui i tagli alle risorse di enti pubblici e ai privati stanno mettendo in ginocchio la nostra economia e comportano lacrime e sangue - come si suol dire - per coloro che hanno di meno, è opportuno dilapidare risorse in spese quali quelle necessarie per un cacciabombardiere d'assalto? Non è forse più consono al buon senso e anche alla nostra Carta costituzionale individuare meglio le priorità e assegnare le poche risorse disponibili a settori maggiormente sensibili e più in sofferenza? questa scelta è compito del nostro Parlamento. Ora, è stato interpretato dai più l'intervento recente del Consiglio supremo di difesa come una entrata a gamba tesa sulla vicenda degli F-35. Vero o falso che sia, ritengo, leggi alla mano, che il citato Consiglio non abbia alcun potere specifico in materia. Alla fine della scorsa legislatura, con la legge 31 dicembre 2012, n. 244, dopo ampia e specifica discussione, si era coscientemente e volutamente modificata la normativa in merito, con ampia maggioranza, attribuendo al Parlamento e alle sue competenti Commissioni di merito un potere preciso di intervento e di decisione su determinati programmi del Ministero della difesa, nello specifico sui sistemi d'arma, potere del Parlamento di certo prevalente rispetto alla volontà del potere esecutivo. Giusto o sbagliato che sia, d'accordo o meno che si sia, questa è la legge del dicembre 2012 e le norme che regolamentano attività e competenze del Consiglio supremo di difesa non spostano di una virgola, allo stato, il panorama istituzionale menzionato. Per quanto concerne la mozione che sto illustrando, non posso non rilevarne i numerosi punti di convergenza rispetto alla mozione avente come primo firmatario il senatore Zanda. Non potrebbe essere diversamente, considerato che in entrambe si sostiene la necessità di dare impulso ad una dimensione europea di difesa comune e soprattutto di pieno rispetto delle prerogative del Parlamento previste dall'articolo 4 della legge del 31 dicembre 2012, n. 244. più in particolare al Partito Democratico, il contenuto del programma elettorale del Partito Democratico in proposito, lì dove veniva letteralmente scritto: «Il Partito Democratico condivide la preoccupazione dell'opinione pubblica sulle spese per gli armamenti. Fermo restando che le esigenze di difesa e di sicurezza dello Stato si sono radicalmente modificate, ma restano, bisogna assolutamente rivedere il nostro impegno per gli F-35. La nostra priorità è il lavoro». Il lavoro, in tutte le sue sfaccettature; e perché mai si dovrebbe derogare a questa priorità? Forse per dare spazio a *lobby* industrial-militari, che negli anni passati, ma anche di recente, si sono caratterizzate e sono ricordate soprattutto per storie infinite di tangenti, corruzioni e malaffare, nazionali e internazionali? Per tornare ai testi oggi in discussione, in che cosa consiste la diversità tra le due mozioni testé citate? Semplicemente nel fatto che nella mozione di cui sono primo firmatario si chiede la «sospensione immediata» del programma F-35. Ciò in presenza di spese per gli F-35 già programmate e stanziate per quest'anno (500 milioni di euro), mentre per il 2014 sono programmati 534,4 milioni di euro e per il 2015 ne sono programmati 657. Ciò al fine di completare l'acquisto da subito di due o tre cacciabombardieri d'assalto F-35 e per l'acquisto nei prossimi mesi di altri sette-otto cacciabombardieri. Proprio quello che, nell'immediatezza, si vorrebbe evitare, senza essere presi in giro, decidendo di destinare i risparmi immediati di spesa, oltre che quelli enormi futuri, a reali priorità, economiche e sociali. Signori del Governo, avete solo l'imbarazzo della scelta, se solo aveste a cuore per davvero le sorti del Paese reale. In conclusione, al Ministro della difesa, che pare amante della locuzione vegeziana, poi mutuata dal più celebre Arpinate, «*Si vis pacem, para bellum*», suggerisco una espressione più consona alla nostra era e alla nostra Costituzione: «*Si vis pacem, para pacem*».

la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, che discutiamo oggi, chiede che l'Italia abbandoni in via definitiva il programma JSF per Lo chiediamo perché riteniamo fermamente che si tratti di una spesa inutile, di un elevato e ingiustificato spreco di denaro pubblico, in un momento storico in cui il nostro Paese non è ancora in grado di risalire la china della recessione e di costruire occasioni di lavoro. Prima ancora di entrare nel merito della mozione in oggetto, mi preme fare chiarezza su quanto accaduto nei giorni scorsi. Mi vorrei soffermare soprattutto sulle affermazioni espresse in sede di Consiglio supremo di difesa, organo presieduto dal presidente Napolitano. Il Consiglio supremo di difesa sostiene che, secondo la Costituzione, le decisioni sull'ammodernamento delle Forze armate spettino all'Esecutivo. Credo giovi ricordare in questa sede che, durante il settennato del presidente Cossiga, vennero ridefiniti i poteri e le competenze del Consiglio supremo di difesa. Esso è, infatti, un organo di informazione e di consulenza del Presidente della Repubblica e, solo indirettamente, del Governo. Visto dunque il ruolo, non sembrerebbe proprio competente a imporre veti alle Camere. Nel testo della delibera del Consiglio si legge che, trattandosi di decisioni operative e provvedimenti tecnici, la competenza specifica per decidere l'acquisto degli F-35 spetterebbe proprio al Governo. Fatta salva detta prerogativa, tuttavia, ad opinione del Movimento 5 Stelle, la situazione deve volgere in altro modo. Se è pur vera la competenza dell'Esecutivo in merito all'attuazione di programmi già approvati dal Parlamento, è impensabile che, all'interno di una Repubblica retta da una forma di Governo parlamentare, il Parlamento medesimo non possa insindacabilmente indirizzare l'attività dell'Esecutivo. Quanto affermato comporterebbe dunque una profonda distorsione del meccanismo istituzionale. In questo modo, si concede un privilegio eccessivo al Governo, ossia quello di rendere le sue decisioni indiscutibili. E questo, in una Repubblica parlamentare, non è accettabile. È assolutamente legittimo che il Parlamento valuti piani pluriennali: quello stesso Parlamento al quale la nostra Costituzione ha riservato un ruolo centrale, rappresentativo e di indirizzo, e non di un organo preposto alla sola ratifica di provvedimenti già presi dal Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Tornando alla mozione in discussione, è necessario sottolineare le criticità emerse nel corso del programma, sono molteplici ed evidenti, già evidenziate dalla collega De Petris. I dubbi inerenti a questo progetto sono sempre crescenti, al punto che molti dei Paesi *partner* hanno fatto un passo indietro. La Gran Bretagna deciderà il numero degli aerei da acquistare dopo la pubblicazione del *Defence and security review* l'Olanda ha avviato un'inchiesta parlamentare a seguito di un pesante voto contrario al progetto; l'Australia non userà gli F-35 come piattaforma esclusiva, acquistando anche altri aerei; la Turchia ha rinviato l'acquisto dei primi F-35; la Norvegia ha minacciato di ripensare le sue scelte sul JSF; la Danimarca ha riaperto la gara per decidere entro il 2015 di quale aereo dotarsi e il Canada ha sospeso la gara per l'acquisto del nuovo caccia. In Canada, in particolare, il ripensamento nasce dalle polemiche scaturite dalle omissioni del Governo sui costi: uno studio indipendente della KPMG ed altri organi di controllo pubblici hanno infatti stabilito che il costo complessivo in 40 anni, includendo anche l'uso e la manutenzione, è di oltre 45 miliardi di dollari, che al cambio attuale sono 33 miliardi di euro

I cacciabombardieri F-35 comportano una spesa esorbitante per il nostro Paese (ben 14 miliardi di euro). È una scelta assai discutibile, per le caratteristiche proprie dell'aereo, adatto per funzioni di attacco in teatri di guerra ed abile a trasportare ordigni nucleari. Nel 2011 c'è stato un *referendum* per porre la parola fine al nucleare come sistema di approvvigionamento energetico, ma continuiamo a mantenerlo nel nostro Paese, perché noi siamo per la pace.

Forse qualcuno non gli ha detto che l'F-22 non era capace di portare nella stiva le bombe B61 che piacciono tanto agli americani e devono piacere per forza anche a noi? Si tratta di una vera e propria arma da guerra. Lo scorso 26 giugno le Commissioni difesa di Camera e Senato, in seduta congiunta, hanno audito il capo di stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Pasquale Preziosa, il quale, durante l'audizione, ha affermato che l'F-35 non è un aereo da combattimento. Infatti, non lo è. Secondo noi è un vero e proprio aereo da bombardamento. Si tratta, insomma, di velivoli atti ad essere impiegati in scenari di guerra, quella stessa guerra che la nostra Costituzione ripudia. Abbiamo forse dimenticato l'articolo 11 della Carta fondamentale della nostra Repubblica: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Forse sganciando qualche bomba nucleare risolveremo le questioni. I nostri Padri costituenti hanno usato il verbo «ripudiare», che racchiude tutta la ripugnanza morale verso gli orrori della guerra e della violenza, cristallizzando in un dovere categorico l'obbligo morale, prima ancora che giuridico, di vietare il ricorso alla guerra come strumento di conquista e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Dunque, è lapalissiano come il progetto F-35 sia completamente incoerente con una politica estera e di difesa che dovrebbe perseguire obiettivi di pace, cooperazione e prevenzione dei conflitti. Va inoltre sottolineato che sono in corso studi internazionali che denunciano gravi difetti degli F-35, tanto da configurarne l'inutilizzabilità. Un progetto evidentemente fallimentare, come sottolineano per primi gli stessi americani. Ricordo alcuni studi commissionati dallo stesso Pentagono, come quello della Rand Corporation (società di consulenza militare di fama mondiale), che ha dapprima stroncato il modello a decollo verticale e, più recentemente, quello a decollo convenzionale, rimarcando i difetti di questi velivoli. Noi, per non farci mancare nulla, ne prendiamo un po' sia a decollo tradizionale che a decollo verticale. Viene criticata infatti la scarsa visibilità, l'inefficienza del casco tecnologico e del radar, ma anche l'assetto, l'autonomia di volo, e non solo: è stato documentato che, allo stato, la manutenzione di questi velivoli verrebbe a costare più del 40 per cento rispetto ai caccia attuali (siamo in un periodo di *cost saving,* quindi aumentiamo le spese anche per la manutenzione). Alla luce di quanto appena detto, il segretario alla difesa Robert Gates ha dichiarato che se la Lockheed non risolverà tutti questi problemi entro due anni (l'azienda ha già apportato oltre ottocento modifiche al progetto iniziale), il Governo americano ritirerà la sua richiesta di acquisto. La domanda è spontanea: ma se addirittura gli americani, che hanno lanciato il programma, con il protrarsi di tali circostanze potrebbero decidere di abbandonare il progetto, perché in Italia il Governo nutre ancora dei dubbi? Considerati inoltre i costi del programma, fonte di prestazioni non solo incerte, come appena detto, ma quasi impossibili e assolutamente non corrispondenti alle esigenze difensive italiane, è opportuno sottolineare, a dispetto di quanto continua ad affermare il Governo, probabilmente più vicino alle logiche delle *lobby* della spesa militare che alle reali esigenze del Paese, quanto le ricadute industriali e occupazionali sarebbero lontanissime dalle aspettative. Gli effetti occupazionali del programma sarebbero per l'Italia assai modesti e decisamente lontani da quella previsione della Difesa di circa 10.000 posti di lavoro, che rievoca promesse di berlusconiana memoria. quando, con le stesse risorse, investendole in opere pubbliche e in politiche per l'occupazione, si potrebbero creare moltissimi posti di lavoro in più. È altresì opportuno ricordare che le nostre aziende non trarranno alcun beneficio in termini di ricaduta tecnologica, essendo noi fornitori di seconda fascia. Infatti, non acquistiamo né tecnologie di prodotto né tecnologie di processo. L'assemblaggio e la manutenzione che verranno svolte a Cameri riguarderanno attività di mera esecuzione di processi, senza conferimento di valore aggiunto e senza la possibilità di ricavarne alcun vero *know-how*, del resto fortemente protetto dagli americani. Da cosa sarebbe dunque rappresentata questa occasione irrinunciabile per l'industria italiana? Mi avvio a concludere. Crediamo dunque doveroso domandarsi: perché il Governo dovrebbe spendere questa esorbitante quantità di denaro pubblico (ribadisco che si tratta di 14 miliardi di euro) per comprare degli aerei da guerra quando abbiamo un Paese investito da una crisi economica devastante? È uno spreco che assolutamente non possiamo permetterci. *(Applausi dal Gruppo* *M5S).* In un momento di profonda recessione, come quello che stiamo vivendo, non si può non riflettere su quali siano le priorità del Paese: non sono di certo gli F-35. Il problema della disoccupazione è una priorità; rilanciare l'economia è una priorità. È chiaro dunque come un Governo degno di questo nome debba dire no, senza se e senza ma, a una simile follia. Colgo l'occasione per ringraziare l'associazione Avaaz, che sul suo sito "www.avaaz.org" ha già raccolto più di 380.000 adesioni. Forse è anche il caso di ascoltare un po' di più i cittadini. Grazie *(PD)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la mozione che abbiamo presentato e ci apprestiamo a discutere oggi riguarda un tema di assoluta rilevanza, relativo al nostro sistema di difesa e sicurezza nazionale. È un tema su cui il Parlamento ha una responsabilità primaria, sia pure in interazione con il Governo: ha la responsabilità di fissare gli indirizzi, le finalità, le priorità, le linee di sviluppo che intendiamo assegnare al nostro strumento militare, sia sul territorio nazionale che nel contesto internazionale; ha altresì la responsabilità di verificare la compatibilità dei sistemi d'arma nel quadro degli indirizzi generali. una serie di questioni delicate ed importanti che attribuiscono al Parlamento una maggiore responsabilità nel valutare con scrupolo e attenzione congruità e coerenza delle scelte, per le quali si rendono necessarie valutazioni e approfondimenti specifici che consentano al Parlamento stesso di esercitare una vera espressione di merito, non solo quindi dichiarazioni di principio. Discutiamo una mozione, un atto di indirizzo che ovviamente non può che esprimere alcune direttive, indicare alcune necessità e, come la mozione che stiamo esaminando, introdurre uno strumento di approfondimento. Il dibattito di oggi può evidentemente solo accennare un argomento estremamente complesso che richiederebbe ben altra analisi. È senz'altro positivo, però, che il Parlamento si soffermi sul punto di evoluzione del nostro strumento militare e faccia una sorta di ricognizione, ribadendo la centralità del Parlamento su questi temi, partendo dalla questione relativa al programma degli F-35, con un approfondimento che richiede impegno e tempo per esaminare in profondità tutti gli elementi del sistema e del suo equilibrio. Questo rappresenta il testo della mozione che discutiamo oggi. Tale testo rappresenta un punto di equilibrio, individuato alla Camera e che i Gruppi proponenti hanno ritenuto opportuno ribadire negli stessi termini al Senato, sugli orientamenti del nostro strumento militare, sulla direzione da imprimere al nostro sistema di difesa e sulla verifica del progetto di acquisizione del sistema d'arma degli F-35; verifica che, evidentemente, non può essere effettuata se non nel contesto di un'analisi più ampia. In questo senso, il testo non poteva che partire dalle coordinate della nostra Costituzione, il già articolo 11 innanzitutto, che esplicita il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come criterio per risolvere le controversie internazionali. Il secondo periodo dello stesso articolo 11 esplicita anche un impegno per il nostro Paese a contribuire a creare un ordine internazionale basato sulla pace e la convivenza democratica a sostegno in particolare dei popoli più oppressi e, quindi, ad essere un soggetto attivo nell'ambito delle organizzazioni multilaterali sullo scenario internazionale. Vi è poi l'articolo 52, la cui applicazione ha avuto un'importanza storica nel far evolvere il senso di appartenenza alla comunità e che in sostanza ha impresso un'accelerazione alla nozione di impegno civile.

Oggi che la crisi economica e i mutamenti dello scenario geopolitico stanno determinando un'accelerazione sull'integrazione della difesa europea, noi dobbiamo iscrivere il nostro progetto di difesa e sicurezza nazionale nel più generale disegno di difesa dell'Unione europea, nella consapevolezza che non è in discussione, come impone la nostra Costituzione, la partecipazione del nostro Paese alla generale assunzione di responsabilità della comunità internazionale per la difesa della pace e della sicurezza. In questo senso va il riferimento al prossimo appuntamento del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre prossimi; il processo di integrazione della difesa europea che, in passato, ha difettato di strategia e di coerenza, oggi appare con tutta evidenza indispensabile per permettere all'Unione europea di svolgere un ruolo a favore della sicurezza e della stabilità internazionale e, tramite lo sviluppo di una base comune industriale e tecnologica, per la stessa crescita economica e la competitività dell'Unione. L'importanza dell'appuntamento di dicembre è, tra l'altro, confermata dal fatto che le Commissioni 4a e 14a del Senato hanno già iniziato un approfondimento sul prossimo Consiglio europeo di dicembre, che intende coinvolgere il Parlamento sulle tematiche in questione e costituire uno stimolo al Governo ad assumere la priorità di rilanciare il processo di integrazione europea su difesa e sicurezza e a promuovere attivamente lo sviluppo di programmi comuni europei. Il tutto mentre la Difesa sta procedendo ad una continua riduzione del proprio bilancio. È ovviamente comprensibile che nell'attuale contesto economico anche il settore della difesa debba responsabilmente fare la propria parte. Il punto è che la nostra Difesa ha già avviato il percorso di razionalizzazione e riqualificazione della spesa militare delineato dalla legge n. 244 del 2012, che rappresenta una vera e propria riforma di sistema. Questo è il punto in cui si trova la nostra Difesa in sintesi: la necessità di bilanciare le capacità operative con le risorse disponibili. A giudicare da alcune posizioni espresse anche in quest'Aula sull'argomento, si direbbe che oggi il nostro Paese stia La realtà è esattamente all'opposto. Vi è una esigenza di ammodernamento degli strumenti operativi, che sono ormai a fine vita operativa, ma, come riportato anche da un autorevole centro di ricerca indipendente, il dato di fondo, non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa (e sottolineo in particolare per il nostro Paese, come indicato nella mozione che stiamo discutendo), è una lenta ma costante erosione complessiva dei bilanci della Difesa; un processo inevitabile vista la grave crisi economica e finanziaria. Tuttavia, c'è anche un altro aspetto del problema: la nostra partecipazione attiva alle iniziative allo sforzo collettivo della comunità internazionale per la pace e la stabilità, non può essere data per scontata senza dotarsi di efficienti strumenti operativi e di politiche che riescano a prevenire i conflitti prima della fase violenta. Penso che le agende dei Paesi occidentali debbano integrare strumenti preventivi di gestione dei conflitti agendo con forza sul dialogo, con la diplomazia, stato detto, di *peace keeping* e di *intelligence*, ma è chiaro che per costruire la pace e per parlare di confronto, di partecipazione, di condivisione di programmi e di progetti europei ed internazionali, bisogna, cari colleghi parlare con coraggio, obbligatoriamente, di efficienti strumenti operativi e cautelativi. Abbiamo quindi la necessità di procedere all'ammodernamento del nostro strumento militare, che rientra, come dicevo, nel processo di razionalizzazione delle spese in corso. Dobbiamo continuamente alimentare il nostro impegno, per essere credibili e concorrere alla stabilità internazionale, con un ruolo coerente con le aspettative di un Paese moderno e pienamente coinvolto nella politica di sicurezza europea e dell'Alleanza atlantica. Ora, in conclusione, sono chiare due cose: la prima, è la centralità del Parlamento; la seconda è che lo strumento dell'indagine conoscitiva sarà utile ad approfondire e a verificare, prima di una espressione di merito, gli aspetti tecnici ed economici, in ordine anche agli aspetti quantitativi e qualitativi e di strategia industriale del programma F-35 che sono emersi nel dibattito in corso. Ribadisco, a conclusione del mio intervento, che un'indagine conoscitiva condotta dal Parlamento in merito alle prospettive strategiche del nostro sistema di difesa, sulla sua sicurezza e quindi anche in merito ai sistemi d'arma da adottare (in particolare sul punto degli F-35), tenuto conto della presente situazione economica, delle alleanze in cui ci collochiamo, delle connesse esigenze di interoperabilità e delle ricadute occupazionali che dalle diverse opzioni possano conseguire, rappresenta la migliore soluzione e di buon senso.

programma pensato e progettato negli Stati Uniti, con un coinvolgimento di altri otto Paesi. Anche sugli F-35 c'è un'attenzione molto forte da parte del mondo organizzato della società civile,

ma, attenzione, non sono mancate voci critiche da una parte degli stessi settori militari, italiani e internazionali. Ecco perché un atteggiamento critico sugli F-35 non va «abbattuto»; ecco perché gli F-35 devono chiedere alla politica un salto di qualità: cultura progettuale, lealtà e correttezza di informazione, capacità di scegliere la strada migliore. Alla Camera si è giunti ad un primo risultato, quello di non procedere senza che il Parlamento si sia espresso nel merito; si è così recepita concretamente concretamente la legge n. 244 del 2012, che per la prima volta sposta la decisione, coinvolgendo i due rami del Parlamento, come avviene nelle democrazie più avanzate e mature. Adesso qui da noi, al Senato, si sta facendo lo stesso percorso, ma ci viene chiesto di fare di più in ordine a tre punti critici molto diffusi e condivisi. Il programma non è mai stato discusso a sufficienza in Parlamento, è quindi necessario avere più tempo per approfondire, conoscere e valutare meglio. Ci sono dubbi molto forti sulla qualità tecnica degli aerei, tanto che il Pentagono e gli stessi tecnici che hanno lavorato al progetto hanno espresso in diverse occasioni perplessità e perfino la produzione è stata più volte interrotta. I costi di partecipazione al programma sono lievitati e oggi risultano troppo elevati. Un paese serio, attraversato da una crisi senza precedenti, deve interrogarsi sulla necessità di spendere ben oltre 14 miliardi di euro per l'acquisto di una specifica arma di offesa. C'è un aspetto che deve essere preso in seria considerazione e che avanza una critica strutturale al programma F-35: l'Europa è esclusa da tale progetto, anzi si può senz'altro sostenere che il progetto si è posto al di fuori della necessità di costruire un modello integrato Sono sempre più convinto che occorra costruire gli Stati Uniti d'Europa nei vari campi della politica, del sistema finanziario fiscale, dell'università, della ricerca, della cultura e della solidarietà. Anche chi è cresciuto nella cultura della pace, come me, non può voltare le spalle alla necessità di creare un inedito moderno modello di difesa europeo. Non è da escludere che un modello integrato europeo potrebbe conciliare le due urgenti necessità: abbattere di molto i costi degli armamenti e avere una difesa europea moderna e tecnologicamente avanzata. I sostenitori del programma degli F-35 hanno spesso utilizzato il tema della ricaduta produttiva ed occupazionale sulla nostra economia e su alcuni particolari territori, problema non da poco, ma si è scoperto che tale ricaduta è stata spesso enfatizzata e strumentalizzata. I risultati sono molto al di sotto di quelli annunciati, quindi è necessario anche in questo caso assumere un atteggiamento più critico è meglio informato. Mettere in discussione quindi il F-35 non è da irresponsabili o da semplici cultori del disarmo; può diventare una necessità seria e fondata. Abbiamo bisogno di una sostanziale sospensione per decidere in tempi brevi quale modello europeo di difesa e di quali sistemi d'arma dobbiamo fruire in un contesto di riduzione della spesa militare, al fine di rilanciare l'Italia e l'Europa dei diritti e del lavoro produttivo in settori civili ed ecosostenibili. Certo, in questi anni sono stati fatti passi in avanti sulla riduzione della spesa militare.

Per questo è giunto il momento per il Parlamento di valutare meglio, bloccare questo programma e fare in modo che il nostro Paese stia in Europa a testa alta, con un modello di difesa più adeguato e con risorse da destinare, in questo momento di crisi, a settori civili così importanti per il futuro della crescita e occupazionale dei nostri giovani.

vari punti: il bilancio del nostro Paese colpito duramente dalla crisi economica, questioni etiche legate al tema della pace e il ruolo strategico che l'Italia può svolgere all'interno dell'Unione europea. noto a tutti che noi di Sinistra Ecologia e Libertà siamo da sempre contrari a questo progetto e siamo per fermarlo immediatamente. Gli F-35, è stato già detto, sono strumenti bellici offensivi, aerei di attacco in piena contraddizione con l'articolo 11 della Costituzione. Noi siamo pacifisti e crediamo che ogni euro speso in armamenti sottragga risorse alla spesa sociale: si tratta di un enorme spreco di risorse pubbliche che andrebbero investite per rilanciare l'economia e il lavoro. La nonviolenza come mezzo di risoluzione dei conflitti personali che abbiamo praticato in questi anni fa parte della nostra identità e l'abbiamo praticata nelle nostre relazioni personali e familiari, nel nostro modo di discutere e nella lettura che abbiamo dato dei processi d'involuzione della nostra società, società, oltre che nelle tante marce per la pace cui abbiamo partecipato come laici insieme a tanti credenti. Con il costo di un F-35, come è stato detto, potremmo mettere in sicurezza 285 scuole italiane, prevedere indennità di disoccupazione per 17.200 lavoratori precari, oppure creare ben 3.500 nuovi posti di lavoro attraverso la costruzione di 387 asili nido, asili nido, garantendo la copertura a 11.610 famiglie! Atti concreti dunque, molto importanti nell'epoca del decreto del fare. Veniamo tacciati di pacifismo ideologico, ma non abbiamo remore a confrontarci anche sulla validità dell'operazione in un'ottica di politica industriale e di ruolo dell'Italia a livello internazionale: in entrambi i casi, quella degli F-35 resta un'operazione sbagliata. Gli F-35 sono inutili, troppo costosi, ad oggi inaffidabili (come tanti studi ci dicono), senza vantaggi tecnologici né ricadute occupazionali significative; investimenti faraonici che costeranno al nostro Paese ben 14 miliardi di euro soltanto per l'acquisto dei caccia e 52 miliardi per la gestione a pieno regime; tutto questo avviene mentre il presidente Letta considera una vittoria strategica lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per il lavoro dei giovani. È uno schiaffo alla nostra partecipazione passata al progetto Eurofighter, i cui aerei costano peraltro la metà e hanno caratteristiche tecniche superiori anche in termini di affidabilità; è un progetto che garantisce un ritorno economico e tecnologico e sono già in uso nell'esercito italiano in nome della costruzione di un sistema di difesa europeo. Si tratta di un progetto passivo con poche ricadute in ambito occupazionale. I mille nuovi addetti di cui alla fine si parla non sono di nuova occupazione, ma derivano dallo spostamento degli addetti previsti oggi dal progetto Alenia-Eurofighier, lasciando competenze, ricerca e la vera ricaduta occupazionale altrove. In questi anni è stata la riconversione delle imprese belliche ad avere una vera ricaduta occupazionale. Alla fine degli anni Ottanta si usarono

controllata dalla danese Vestas, è nata da un progetto di riconversione militare di Alenia, la ex Aeritalia, ed anche che la Oerlikon Graziano, che produce a Bari sistemi di cambi per auto di lusso e per trattori, è nata dalla diversificazione verso l'uso civile di Oto Melara; e ancora: gli aerei civili di Agusta, gli *yacht* di Fincantieri. La riconversione dell'industria bellica è non soltanto possibile, ma fornisce grandi opportunità di lavoro, soprattutto in questo momento in cui la crisi economica porta con sé una positiva riduzione della spesa militare. pare aver dato l'avallo al progetto di Pansa di rivedere il settore civile di Finmeccanica, che invece sarebbe da potenziare e sviluppare. Noi diciamo al Governo che non è dismettendo in questo momento il settore civile che si può favorire la ripresa e rilanciare l'occupazione. A dirigere Finmeccanica servirebbe una personalità proveniente dal mondo industriale dell'alta tecnologia, un *manager* capace ed innovativo, in grado di integrare e sviluppare in ambito civile i settori più avanzati. Invece si sceglie De Gennaro, un alto dirigente della polizia, di cui riconosciamo i meriti da investigatore ma i demeriti per la gestione fallimentare dell'ordine pubblico al G8 di Genova: è anche politicamente sua la responsabilità della macelleria cilena avvenuta alla Arriviamo a un ultimo punto che ci sta a cuore: la sudditanza dell'Italia ad un Paese amico come gli Stati Uniti, la migliore dimostrazione di che strana idea di Europa ha in mente la maggioranza delle larghe intese. Un elemento grave della vicenda F-35 riguarda il ruolo che il nostro Paese vuole giocare nell'Unione europea e nello scacchiere mondiale. Molti di noi appartengono ad una generazione che non è stata antiamericana, ma proprio per questo non sentiamo la necessità di dimostrare di non esserlo più assumendo posizioni di sudditanza verso gli Stati Uniti. Siamo una generazione che appartiene profondamente all'Europa, che considera i Paesi europei non come alleati ma come compagni di viaggio, i propri abitanti concittadini, e insieme agli altri Paesi europei ci consideriamo alleati degli Stati Uniti. È per questo che riteniamo che il progetto degli F-35 è completamente sbagliato, frutto di un'impostazione di politica estera cosiddetta del doppio forno. La vicenda degli F-35 dimostra l'incapacità di una generazione di politici e militari che ha affossato dunque le potenzialità tecnologiche del nostro Paese, facendone pagare il conto ai cittadini. La ministra Bonino, con la quale siamo in disaccordo totale sulla vicenda Snowden, sostiene che in Europa abbiamo 27 eserciti inutili e costosi: due milioni di persone in divisa, magari neppure dialoganti tra loro. Ecco, è necessario quantomeno costruire un esercito unico europeo, rivedere le dislocazioni dei militari nel territorio italiano, far dialogare e mettere in comune le esperienze, ridurre di gran lunga le spese, le sovrapposizioni e gli sprechi; questo può e deve essere fatto oggi: non è necessario attendere la nascita dell'Europa federale, che anche noi di SEL auspichiamo particolarmente. In campagna elettorale i programmi del centrosinistra, quelli di Italia Bene Comune, erano molto chiari sugli F-35 e non capiamo, o forse la capiamo molto bene, questa improvvisa timidezza del Partito Democratico. Ai cittadini italiani il taglio degli sprechi e delle sovrapposizioni lo dobbiamo. Possiamo uscire da questa crisi economica soltanto con un'accelerazione ed un rafforzamento del percorso di integrazione europea, per abbandonare l'Europa dei tecnocrati e della sola *austerity*, nata nella teste soprattutto delle banche, non dei nostri cittadini. Oggi ci assumiamo una grande responsabilità nei confronti degli italiani: oggi decidiamo se investire risorse contro la povertà o se invece comprare aerei che possono lanciare armi atomiche. Andate a spiegare allora ai cassaintegrati, ai disoccupati, ai giovani precari che è più giusta questa seconda opzione. Questa decisione spetta tutta al Parlamento italiano e consideriamo molto grave che il Consiglio supremo di difesa, presieduto dal presidente Napolitano, abbia sostenuto che il Parlamento non può porre veti all'adesione al progetto. Serve allora una vera rivoluzione culturale; bisogna decidere da che parte stare. Noi siamo per l'Europa, per la pace, per uno sviluppo compatibile, per l'Italia bene comune. Noi non ci renderemo complici, mai, nemmeno indirettamente, di orrori di guerra.

il mio intervento come rappresentante del territorio novarese, che accoglie, nell'ambito dell'aeroporto dell'Aeronautica militare di Cameri, la FACO, quale centro di assemblaggio, vuole porre subito in evidenza come il programma F-35 non abbia portato finora ricadute occupazionali ed economiche sul nostro territorio. previsioni iperboliche tanto sbandierate negli anni passati (la «panacea occupazionale» del novarese) si sono rivelate infatti un'ennesima illusione. I dati in merito all'occupazione ci mettono di fronte ad una situazione ben diversa da quella che era stata promessa i posti di lavoro deriverebbero per la gran parte da mobilità di occupati sovrannumerari dell'Alenia di Torino o di altri comparti di Finmeccanica. I nostri concittadini, che hanno subito una forte contrazione occupazionale in tutti i settori e hanno quindi a maggior ragione sperato nei 15.000-20.000 posti di lavoro promessi, si sentono ingannati, perché questi sono andati sempre più a scalare negli anni e oggi sono ridotti a meno di un decimo (secondo i dati più ottimistici). Ribadisco, perché sia chiaro: i nuovi posti di lavoro alla FACO di Cameri ammonterebbero solo a qualche centinaio, e le ricadute occupazionali locali sarebbero minime. Nel corso degli ultimi due anni e mezzo il Partito Democratico di Novara, attraverso una commissione specifica, ha ascoltato e discusso con centinaia di cittadini - questi, al contrario, sempre più numerosi! - ed ha incontrato i principali attori del territorio, così come esperti ed esponenti di carattere nazionale. È stato approvato unanimemente un documento che raccoglie le più evidenti criticità del programma F-35, circa la sostenibilità dei costi (di acquisto e di gestione), la validità del sistema d'arma e la sua rispondenza alle esigenze di difesa nazionali ed europee, e chiede una corretta e realistica riflessione sulle ricadute tecnologiche, industriali e - come ho già detto - occupazionali sull'Italia e sull'Europa. II balletto dei numeri sui costi e sulla quantità dei caccia F-35 che l'Italia acquisterebbe è stato elemento di grande disorientamento. Facciamo il punto: ad oggi, l'Italia si è impegnata ad acquistare 11 velivoli, se i dati sono corretti; circa 2 miliardi è costata la fase di ricerca, svolta negli Stati Uniti, e ogni cacciabombardiere costerebbe circa 150 milioni di dollari (naturalmente con le dovute La mozione Zanda e altri impegna il Governo a non procedere a nessuna fase di ulteriore acquisizione finché il Parlamento non si esprima nel merito. Riteniamo fondamentale, per il presente e il futuro della politica di difesa, la norma che più volte viene richiamata nella premessa e nel dispositivo della mozione: la legge 31 dicembre 2012, n. 244, che attribuisce la competenza in merito al futuro della commessa militare in capo al Parlamento. Il merito di questo risultato - come ha detto il senatore Casson - è in particolare del PD, che qualche mese fa ha voluto imporre questa norma. Solo qualche mese fa si è deciso di non transigere con queste chiare motivazioni: la coerenza dell'adozione dei programmi del sistema d'arma a seguito di valutazioni riguardanti la situazione geopolitica internazionale, l'individuazione delle sfide strategiche incombenti, la coerenza e la congruità degli investimenti militari, che devono essere contestualizzati alla luce delle condizioni generali della finanza pubblica e della crisi economica e sociale che il nostro Paese sta attraversando. Tutto ciò deve essere in capo al Parlamento. Oggi, con la mozione Zanda, riteniamo venga data una significativa risposta anche al territorio novarese, che da anni chiede verità su questo programma e che mette a sua volta a disposizione le competenze acquisite, ritenendo di vantare un credito di ascolto. Ringraziamo a tal proposito i parlamentari che nel corso degli anni hanno seguito da vicino l'argomento nelle Commissioni competenti e mantenuto i contatti con il nostro territorio. A fronte di un movimentismo e di una crescente contrarietà dell'opinione pubblica rispetto al programma F-35, lo sforzo del nostro partito, che è un partito di Governo, è l'argomentazione di merito, la costante ricerca dei dati reali. Al di là dei problemi tecnici, riteniamo che la mancanza di sovranità tecnologica del velivolo sia un tema di grandissima rilevanza. Quindi, rispetto ad altri programmi europei che peraltro contribuirebbero a rafforzare una linea di difesa della Comunità europea, la scelta degli F-35 è davvero produttiva sul piano economico ed industriale italiano ed europeo? È quanto mai opportuno e doveroso che il Parlamento italiano affronti questi temi con l'obiettivo di verificare il programma F-35 in un'ottica di sviluppo della dimensione di difesa europea auspicata nella mozione presentata

Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, non vorrei soffermarmi molto sulle considerazioni tecniche emerse in questi giorni dalla stampa e dall'informazione. Proviamo ad immaginare per un attimo una situazione di guerra in cui venissero impiegati davvero gli F-35. Tale ipotetico scenario, peraltro, dovrebbe difficilmente verificarsi se rispettassimo l'articolo 11 della nostra Costituzione. Supponiamo, comunque, che in un momento di difficoltà arrivino i nostri F-35 a salvare la situazione. Attenzione, però: facciamo la guerra solo se il tempo è bello perché con l'umidità ci sarebbero problemi di decollo e di atterraggio. Anzi, facciamola con il tempo bello e con una temperatura non troppo elevata, se vogliamo essere sicuri che i nostri aerei non incontrino difficoltà aggiuntive. Anzi ancora, facciamola solo contro aerei simili ai nostri perché tutti gli altri modelli potrebbero abbatterci con troppa semplicità. Tutto ciò non è logico. Tutto ciò è ridicolo. Ma la guerra non è ridicola: la guerra è orribile, è illogica. Ricordiamolo. Queste scelte sono per noi prive di senso e lo sono sin dalla decisione iniziale di aderire ad un programma tecnicamente opinabile e che pare metta in pericolo gli stessi piloti: i nostri figli, i figli della Patria. Ma le vite umane sono considerate calcolate? Dove? Nella voce «costi» o nella voce «imprevisti prevedibili»? Un progetto frutto di chissà quali idee ed accordi economici non accettabili, di costi esagerati ed inopportuni in questo periodo di totale crisi strutturale. Un progetto poco conveniente persino dal punto di vista del ritorno economico e tecnologico in collaborazione con il principale *competitor* dello stesso settore. Il 26 giugno scorso, la Camera dei deputati ha approvato una mozione rivolta al controllo rigoroso del progetto, ma senza il coraggio di interrompere definitivamente l'operazione con la prerogative di «non procedere a nessuna fase di ulteriore acquisizione senza che il Parlamento si sia espresso nel merito, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244 ». Parliamo di assenza di coraggio perché nelle vostre mozioni troviamo utilizzati i termini «sospendere», «ridefinire», «in tempi rapidi»: tutti formulazioni dai confini imprecisi e incerti nei modi e nei tempi. I termini che vorremmo trovare dovrebbero invece essere: «fermare», «interrompere», «chiudere», «definitivamente». Signori miei, questo non è il Governo del fare, questo è il Governo del prorogare, differire, posticipare, rinviare, procrastinare. Basta! Coraggio, miei senatori, abbiate il coraggio di rinnovarvi, abbiate il coraggio di cambiare rotta! Come se ciò non bastasse, nella seduta del 3 luglio il Consiglio supremo di difesa, che non è altro che un organo di informazione e consulenza e consulenza del Presidente della Repubblica, si è espresso attribuendo al Governo la responsabilità delle decisioni in merito alla questione. Si tratta, secondo noi, dell'ennesimo svilimento delle prerogative del Parlamento, delegittimato nelle proprie scelte Cari colleghi, perché non siete quanto meno irritati? Non era forse nella vostra mozione la volontà di sospendere o interrompere immediatamente la partecipazione italiana al programma? Sogno o son desta? Siamo ancora in una Repubblica? In una Repubblica parlamentare? Non è forse il Parlamento ad essere sovrano, visto il ruolo centrale attribuitogli dalla nostra Costituzione? Non vorrei, miei colleghi, che ci fossimo tutti arresi e autorelegati a un ruolo subalterno. Tutto ciò non è logico. È inammissibile. Il nuovo modello di difesa, nonostante l'abolizione della coscrizione obbligatoria e la riduzione degli effettivi e delle strutture, ha comportato una crescita delle spese militari in questi due decenni. *(Applausi dal Gruppo A fronte di tagli pesanti a istruzione, università e sanità, quella militare è l'unica spesa pubblica a crescere costantemente. In questi due decenni il risparmio per i tagli al personale è stato stornato in nuovi e costosissimi sistemi d'arma. Per questo riteniamo necessario arrivare - come hanno fatto gli altri Paesi della NATO, quali il Canada e la Gran Bretagna - alla revisione del programma di acquisto relativo agli F-35, troppo costosi e incompatibili con la vocazione di pace che dovrebbe avere il nostro Paese. Coraggio, miei senatori: abbiate il coraggio di attuare il cambiamento che il Paese vi chiede! Noi siamo chiamati a una scelta, a un atto di discernimento. Il discernimento deve essere attuato considerando tutte le alternative generate dalle condizioni al contorno. Vogliamo o no ammettere che il contesto degli ultimi quindici anni è cambiato? Allora, in qualunque problema complesso, dove le condizioni al contorno cambiano, cambiano anche le soluzioni. Le soluzioni di allora non devono più essere le stesse di adesso, non possono! Pertanto, con la mozione del Movimento 5 Stelle vi chiediamo non di cambiare le idee, non di fare passi indietro, ma di valutare che la situazione nel suo complesso è cambiata e, quindi, è cambiata anche la sua soluzione. Non possiamo spendere 13 miliardi di euro per l'acquisto di questi velivoli quando in Italia quasi la metà degli edifici scolastici non possiede le certificazioni di agibilità per cento non ha il certificato di prevenzione incendi e il 36 per cento degli edifici ha bisogno di interventi di manutenzione urgenti. Tutto ciò non è logico. È sconcertante. L'Italia di oggi non ha il problema di scegliere le vacanze. Le famiglie hanno il problema del lavoro. I padri di famiglia non riescono a mantenere i propri figli. L'Italia è ormai vicina al punto di non ritorno. Se vogliamo le armi, allora usiamo quelle che Nelson Mandela consiglia:

per richiamare un epiteto poco elegante rivolto al nostro Gruppo solo pochi giorni fa da un rappresentante del Governo. Mi riferisco alla deficienza in senso semantico. «deficere» etimologicamente, dal latino, significa mancare di qualcosa, essere mancanti. Ebbene, questo essere deficienti può essere nel nostro caso un'opportunità, un modo nuovo e non ipocrita di affrontare le questioni fondamentali, scevri da ogni retaggio e condizionamento. Siamo cittadini non avvezzi all'usuale commistione tra affari e politica, e ne andiamo orgogliosi. Questa mancanza per noi non è un *handicap*, è un essere diversamente abili *(Applausi dal Gruppo M5S)* nella comprensione e nell'analisi dei meccanismi che ci tengono lontani da un mondo cieco e sordo dinanzi alle vere necessità degli italiani. Non siamo deficienti: il termine giusto è nuovi, rinnovatori, per una Repubblica dei cittadini e non per una Repubblica dei saggi consulenti, troppo spesso relegati all'uso surrogato e improprio del potere che spetta al Parlamento. Ecco chi siamo noi.

Ecco chi siamo noi. Noi cerchiamo i nostri interessi negli interessi di tutti e non gli interessi di tutti nei nostri interessi. Ecco qui dove sta la deficienza vera: sta in un Parlamento mancante e quindi deficitario nelle proprie prerogative istituzionali e democratiche, solo dedito all'approvazione degli atti di un Governo altrettanto deficitario e dedito al mantenimento statico di un equilibrio politico im-pos-si-bi-le, come testimoniato dalla modalità con cui il Parlamento ha sinora affrontato la questione della riduzione degli armamenti e dalla singolare risposta del Governo. Vorrei sottolineare che questa non è un'Assemblea di deficienti, ma è sicuramente un'Assemblea deficiente, sempre in senso semantico. *Melius abundare quam deficere*. Signor Presidente, termino con un ultimo omaggio rispettoso a Madiba: «La pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare». Anch'io, signor Presidente, nel mio piccolo ho un sogno: il sogno di passare per le strade e di essere indicata non come colei che possiede immunità parlamentare, ma umanità parlamentare.

passando per le strade, rischia di essere insultato per quello: ci insultano per altre cose, questo non è più un insulto corrente. È difficile intervenire in questa discussione, signor Presidente, perché

È molto facile, in una situazione di crisi come quella che vive oggi il nostro Paese, fare una facile equazione: meno aerei, più asili, più lavoro. *(Applausi una mozione parlamentare approvata determinasse questo. Sappiamo tutti che non è così, e dovreste saperlo anche voi. Queste sono scelte che al momento opportuno, eventualmente, passeranno all'interno del bilancio il Senato e la Camera approveranno. Il Gruppo che io, insieme a tanti in quest'Aula, rappresento ha depositato la mozione approvata con una larga maggioranza dalla Camera dei deputati; quella mozione, di fatto, sospende per sei mesi il programma, rimettendo eventuali ulteriori acquisizioni nelle mani del Parlamento, cosa che prima non avveniva. sospendere il programma alla luce di quello che a dicembre si discuterà in sede di Consiglio europeo, ossia rispetto all'avvio - speriamo: per questo ci battiamo e nella nostra mozione c'è un impegno al Governo a operare in questo senso - di un processo di integrazione della difesa a livello europeo. Di questo noi non discutiamo. Non stiamo discutendo di una mozione presentata dalla maggioranza che dichiara guerra a qualche Stato o che aumenta i fondi aumenta i fondi per la difesa o per l'acquisto degli aerei. Anzi: siamo l'unico Stato che negli ultimi nove anni ha diminuito del 19 per cento le Siamo quelli che spendono di meno in Europa. Io penso che dovremmo spendere ancora di meno, e per questo serve la fase di riflessione che noi abbiamo aperto. dipende dalla prosecuzione del processo di integrazione di difesa europea. Tutti noi possiamo essere pacifisti all'eccesso: anch'io sono per la pace, però capisco che quando si governa uno Stato come l'Italia, dentro l'Europa, con quello che noi rappresentiamo sullo scenario europeo e, in particolare, mediterraneo, con tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente e nel Nord Africa, occorre comunque avere un proprio sistema di difesa. Non possiamo ogni volta invocare, quando è necessario, l'aiuto degli altri, salvo poi dire che c'è l'invadenza di chi viene ad aiutarci, in particolare degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America peseranno sempre meno se andrà avanti un processo di integrazione di difesa a livello europeo, al quale noi dobbiamo partecipare. Cari colleghi, sappiamo tutti che non solo l'Italia, ma anche la Francia e la Gran Bretagna, singolarmente i Paesi europei, di fronte alla Cina, alla Russia, agli Stati Uniti

delle quali fanno parte anche i colleghi del Movimento 5 Stelle e di SEL, nelle quali abbiamo avviato un'indagine conoscitiva sul sistema di integrazione di difesa europea per poter dare un contributo al Governo in vista dell'appuntamento di dicembre.

l'Italia dovrà partecipare con le risorse che noi come Paese dovremo mettere, perché non possiamo pretendere che siano gli altri a difenderci. Un Paese deve avere un sistema di difesa, e se è vero, come dite voi, che nella Costituzione c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra, nella Costituzione c'è anche scritto che noi dobbiamo avere un sistema di difesa per difendere la nostra Patria. Il sistema di difesa integrato europeo è l'approdo verso il quale, con l'approvazione della mozione da noi presentata, noi andiamo, per ridurre le spese e per avere sei mesi

sul rapporto sussistente tra l'uso delle armi e la gestione della democrazia e del principio universale della libertà dei popoli. Questa argomentazione non può esimersi dall'investire in pieno l'annoso dibattito che riguarda l'interpretazione giuridica dell'articolo 11 della Costituzione: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;», recita il primo periodo. La corrispondenza logica tra l'utilizzo di armamenti sofisticati e la volontà di offendere o di guerreggiare non credo possa essere suscettibile di diverse interpretazioni: si utilizzano le armi per sovrastare, in un teatro di guerra, dentro o fuori i propri confini territoriali, un eventuale nemico, o incutere terrore, e quindi sotto forma di potenza deterrente. L'adesione sin dal 1996 in poi, concretizzata nel 1998, al programma *Joint Strike Fighter* in condizione di *partnership* secondaria insieme ad altri sette Paesi con le Forze armate statunitensi ci pone in netta contrapposizione con lo spirito dell'articolo sopra citato fin dall'origine dell'accordo stesso. Tuttavia, qualcuno potrebbe obiettare che c'è il secondo periodo dell'articolo 11, che testualmente recita: «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Sarebbe in questo caso utile che qualcuno spiegasse come l'utilizzo di armi che hanno la capacità di portare sulle loro ali dei missili atomici sia in qualche modo conciliabile con la promozione di organizzazioni internazionali che assicurino la pace e la giustizia fra le Nazioni! Una volta esaminata questa premessa di diritto, un nuovo spunto di riflessione, questa volta di merito, ci viene dai vari *report* internazionali militari sull'efficienza e l'affidabilità di tali macchine di morte. Australiani, danesi, turchi, norvegesi, britannici (storicamente non gli ultimi arrivati in fatto di competenze belliche, ed in particolare dell'aviazione militare) hanno esposto, pubblicamente, vulnerabilità e criticità evidenti sull'efficacia e sulla tenuta non solo in battaglia degli F-35, ma anche nei semplici voli di prova e ricognizione (eccessiva catalizzazione ai fulmini, poco spazio per i caschi piloti, motori lenti), decidendo di limitarne la produzione o di sospendere l'adesione al programma in attesa di rilevazioni tecniche più precise. Il Canada ha rinunciato a dare esecuzione al Programma. Lo stesso Pentagono ha rilevato che i costi e i ritardi del Programma forse non giustificano l'ultimazione dello stesso. Mi chiedo perché noi italiani, laddove il dibattito pubblico ed istituzionale si evolve verso l'estinzione o, quanto meno, la limitazione del nostro contributo militare, anche per evidenti motivi ostativi di *spending review*, nei territori di guerra esistenti oltre confine, dovremmo dare piena esecuzione all'accordo sull'acquisto dei velivoli e non decidere di adottare forme alternative al minimo di sospensione o di rivisitazione dello stesso in termini meno esosi e meno aleatori. II terzo ordine dì motivi per i quali mi trovo decisamente contraria all'acquisto dei cacciabombardieri è chiaramente di tipo economico-finanziario. Non ci vuole un acuto economista per comprendere che una spesa pubblica cosi eccessiva per un progetto tanto vago e di impiego così eventuale e remoto possa essere molto più razionalmente convertita in settori o campi maggiormente sensibili, fragili e bisognosi di urgenti interventi infrastrutturali oggi in Italia. Parliamo ogni giorno di occupazione ai minimi storici, territori da riqualificare per renderli sicuri, competitivi nella produzione, nel *welfare* e nel turismo, di tessuti aziendali falliti che necessitano di rilancio, di risorse imprenditoriali e cervelli che vogliono espatriare, enti territoriali, giustizia, sanità e istruzione da riformare, ricerca universitaria da valorizzare. E vogliamo sprecare mezzi notevoli per potenziare gli armamenti? Non convince, del resto, la velleitaria difesa di chi crede ancora nella gara a «Risiko» della guerra o di chi ha interesse affinché si corra in quella direzione. Il dato che Cina, Russia, Iran, Corea del Nord ed altri abbiano esorbitanti ambizioni militari e che investano parti ingenti della loro ricchezza in armamenti di distruzione di massa non fa cambiare idea. Non è di sicuro la paura, ad oggi del tutto infondata (ed in ogni caso poco cambierebbe nel caso contrario, anche con gli F-35), di essere annientati militarmente da questi eserciti a doverci imporre di modificare il nostro criterio progressista e razionalistico di guardare il mondo ed impedirci di sostenere il progetto europeo di un futuro di compartecipazione pacifica tra i popoli. Ben altre sono le molle culturali ed ideologiche che muovono le economie e le strategie espansionistiche che sono alla base delle scelte belliche di questi Paesi. mi dichiaro assolutamente contraria alla partecipazione italiana al Progetto di realizzazione degli aerei

La discussione di oggi rappresenta il doveroso punto di approdo di un confronto su un argomento complesso e delicato allo stesso tempo. Un argomento su cui tensioni e congiunture sembrano essere state abilmente fomentate più per tornaconto politico che per reali esigenze finanziarie. Ma andiamo per ordine. Quanto affrontato nella mozione non si limita all'opportunità o meno di spendere un determinato *budget* per l'acquisto di una dotazione militare. Va più in profondità: afferisce alle responsabilità che ha il nostro Paese, al suo impegno ad essere parte attiva, responsabile e coerente, di un progetto internazionale del quale ha voluto essere, fin dall'inizio, protagonista. Oggi vogliamo e dobbiamo dare priorità a questo. Le strumentalizzazioni pseudopacifiste o di *austerity* esasperata c'entrano poco con la partecipazione italiana al programma di realizzazione degli F-35. Certamente sono anche comprensibili i ragionamenti che molti muovono nella direzione della inopportunità di una così imponente spesa per lo Stato, considerato il momento e le difficoltà finanziarie del Paese. È possibile comprenderne le ragioni, che sono tra l'altro le stesse che hanno condotto ad un ridimensionamento del numero di velivoli da 131 a 90. In questo, però, si fa fatica a cogliere una reale consapevolezza delle conseguenze che potrebbe avere il ritiro dell'Italia dal progetto, non soltanto in termini di credibilità politica internazionale o di coerenza del ma anche e soprattutto di riflessi economici che un eventuale passo indietro potrebbe comportare, per la perdita di commesse per le industrie italiane e per gli oneri, esponenziali, che deriverebbero dal ritiro dal progetto. Ma i critici, nelle loro affermazioni, si mantengono ben distanti dall'affrontare questi aspetti. Noi, però, siamo ben lieti di approfondirli, ragionando nelle opportune sedi circa l'equazione costi-opportunità, che sembra non aver mai trovato spazio nei dibattiti. Forse perché, affrontando un tale ragionamento, verrebbe meno l'articolato castello di euforia demagogica che da mesi - se non da anni - alimenta il fronte dei critici, e che si riversa in maniera incontrollata anche sulla società civile, fomentando rabbia e malumori che al momento sembrano essere davvero poco opportuni. Ma proprio in questo momento, confondere i due livelli - la demagogia e il mantenimento di un impegno - rischia di essere deleterio e poco fattivo per il futuro del Paese: non soltanto perché mancherebbe il rispetto nei confronti dei cittadini, che non sono realmente informati circa le reali dinamiche del progetto e sui suoi aspetti di presunta criticità; ma anche e soprattutto perché si rischia di bloccare le potenzialità economiche, scientifiche e militari che sottendono questo progetto. Additare il programma come incostituzionale pecca di superficialità analitica oltre che di scollamento con una realtà di cui l'Italia ha inteso farsi carico. Proprio come ricordava qualche giorno fa il ministro Mauro, il cuore del problema sta in un interrogativo: è possibile armare le ragioni della pace, ragioni esposte nella nostra Costituzione? Ed è molto probabile che intorno a questo dilemma si siano costruite tutte le fantasticherie che hanno condotto alla discussione di oggi. Dobbiamo ricordare che la pace è anche difesa; la pace è anche deterrenza, soprattutto in uno scenario tentacolare e complesso sotto il profilo geopolitico come quello attuale. Giocare un ruolo propositivo ed attivo nello scenario internazionale, facendosi carico di determinati impegni e mai sottraendosi alle responsabilità che ne derivano, si colloca proprio in questa direzione. E l'Italia non può permettersi, in questa delicata fase, alcun passo indietro, soprattutto se si guarda al progetto della difesa comune europea. Come qualcuno ricordava, nel dicembre 2013 l'Unione europea tornerà a riflettere sul tema della difesa europea e sulla volontà condivisa di dare forma ad un progetto politico costruito intorno ad essa, che ci auguriamo sia più rispondente e, di conseguenza, più efficace in uno scenario che si evolve. E sicuramente, dalla prospettiva di Bruxelles sarà possibile ritornare a ragionare sulla opportunità del programma degli F-35 con un approccio diverso, un approccio che ora non possiamo assolutamente permetterci. Questo perché i tempi non sono maturi. Infatti, è sotto gli occhi di tutti che la politica estera dell'Unione europea non ha la forza per imporsi in un scenario internazionale, e che dunque deve passare attraverso un percorso di costruzione di un nuovo piano di operatività strategica militare che sappia rilanciare il fine ultimo dell'integrazione europea, vale a dire la pace, pensando ad un progetto di esercito comune e di difesa comune, ad esempio. Soltanto ragionando in questa prospettiva possiamo permetterci di superare le critiche demagogiche e superficiali di chi accusa con rabbia il progetto degli F-35. Partendo da queste premesse, appare inderogabile il rinnovamento dello strumento militare nazionale, che consiste anche nell'acquisizione dei nuovi F-35 quali, come è stato ampiamente evidenziato, andranno a sostituire velivoli che sotto il profilo tecnologico e strategico risultano essere poco fattivi anche perché datati. E come è facile immaginare, la loro permanenza potrebbe rappresentare un rischio per i nostri uomini più che un valore aggiunto. Proprio la consapevolezza di questo ha condotto al programma F-35 già alla fine degli anni Novanta, un programma a cui ha inteso aderire un *parterre* di Paesi con l'obiettivo di creare intorno all'avanguardia tecnologica e alla ricerca scientifica nuovi strumenti di difesa e di sicurezza per lo scenario internazionale. Un impegno nobile - permettetemi di dirlo - che fin dalle prime battute aveva la priorità di coniugare le istanze di pace alla ricerca e allo sviluppo, in chiave europea, creando economia e innovazione e rafforzando l'impegno del nostro Paese, dove però sia l'Europa lo scenario di questo rinnovato impegno. È proprio su questo punto che dobbiamo concentrare la nostra attenzione, per far sì che non si parli più di impegno del singolo Stato, ma di impegno europeo, tale da superare le criticità e le speculazioni politiche e sociali dei singoli Paesi, incrementando l'efficacia delle iniziative e delle misure a garanzia della sicurezza della regione. In questa fase di costruzione dell'identità europea della difesa, l'impegno dell'Italia sui fronti caldi, il riconoscimento del valore dei nostri militari e delle forze di sicurezza impegnate attivamente in aree devastate dalla guerra e dal terrorismo, diventano parte di questo progetto, un progetto che merita rispetto e attenzione. Noi vogliamo dare alle nostre Forze armate gli strumenti per garantire la loro sicurezza e non possiamo minimamente pensare di comprometterne la realizzazione in nome di una speculazione demagogica di cui l'Italia *in primis* sarà vittima. Quindi, il futuro del Paese e dell'Europa tutta non può ruotare intorno alla demagogia anti F-35; deve basarsi sulla comprensione, sull'analisi del progetto e sulle possibilità eventuali di modificarlo e monitorarlo nel tempo e nella qualità. Questo è un impegno che la politica deve prendere nei confronti del Paese e del suo ruolo, partendo però sempre della consapevolezza che stiamo costruendo una nuova identità europea. A questo punto sarebbe auspicabile che le voci critiche promuovessero progetti alternativi o proposte di modifica piuttosto che arroccarsi dietro un presunto pacifismo che sa di tempi antichi e c'entra poco con la realtà attuale. Dinanzi alle sfide globali siate concreti. Mettete da parte le frasi ad effetto e le invettive contro le superpotenze, che manco più creano consensi. Pensate a quello che è il futuro dei vostri figli, a quale livello di sicurezza possiamo aspirare e a che strumenti possiamo garantire e poi magari riparliamone insieme, soltanto quando la demagogia spicciola avrà lasciato spazio alla maturità politica. Dinanzi alla tentazione delle posizioni ideologiche, bisogna saper guardare oltre mettendo al centro l'interesse generale e le potenzialità di un futuro non lontano, puntando al progetto della difesa europea attraverso il quale sarà possibile rivedere l'efficacia dello strumento militare italiano e riadeguarlo alle nuove prospettive. e smettiamo di chiamare in causa testimonianze di comodo, in una retorica della politica che a volte si mostra lontana dai fatti. La politica deve avere il coraggio della responsabilità. Chiudo facendo mie le parole di un grande uomo: la pace è un dono da invocare, è un obiettivo da costruire. Grazie razzi o bombe, «il risultato non cambia, Idriss e Ahmad, otto anni in due. È questa in fondo - mi dico - la maledetta realtà della guerra, la sua mostruosità. È tutto qui.

che spiegasse ad Ahmad Froh e a Idriss che è giusto che loro siano conciati così perché una coalizione militare ha deciso di "sconfiggere il terrorismo" bombardando il loro cortile e il mercato». Bombardandolo. Parole di Gino Strada.

Il nostro magnifico articolo 11 della Costituzione non dovrebbe tutelare noi ed il nostro prossimo proprio da queste cose? L'Italia ripudia la guerra. Lo ha già ricordato l'amico Lorenzo, come molti altri. Non ne ripeterò le parole, sottolineo solo le sue osservazioni: ripudiamo la guerra e compriamo cacciabombardieri abilitati a trasportare e a sganciare ordigni nucleari. Che questi argomenti non facciano breccia e non vi convincano ad abbandonare il progetto F-35 ce lo ha insegnato ciò che è successo alla Camera. Allora proviamo a ragionare in soldi: l'unico argomento che per voi è veramente importante. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Come spendereste 14 miliardi di euro se li aveste a disposizione? Ve lo diciamo noi; ce lo ricordate sempre ad ogni proposta. Le scuole sono insicure? Vergognoso, ma mancano i soldi. Creiamo un fondo per le piccole imprese? Non si può. Istituiamo il reddito di cittadinanza? E i soldi dove li troviamo? È un mantra continuo, ormai. Abbandoniamo questo folle progetto subito e i soldi ci saranno. Ma c'è qualcuno che mi sa dire come reagiranno gli altri Stati al nostro *shopping* bellico? Ci avete pensato? O forse è questo il vero obiettivo: scatenare una forsennata corsa all'acquisto di armamenti per favorire la *lobby* dei costruttori? Noi del Movimento 5 Stelle siamo contrari allo spreco di soldi, alla guerra e a questi dannati cacciabombardieri. Votate pure contro la nostra mozione. Spiegherete agli italiani in difficoltà, agli imprenditori che stanno per chiudere le loro imprese, agli artigiani e ai commercianti che purtroppo, per loro, i soldi non ci sono. Un'ultima cosa, Ministro. Lei ha detto una frase che penso passerà alla storia e non so come verrà valutata: «Per amare la pace bisogna armare la pace». Lei ha figli? Provi a mettere una pistola in mano a suo figlio e a dirgli: «Vai a scuola e fai la pace con i tuoi compagni»! Grazie *(PdL)*. Signora Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, negli anni il Parlamento è intervenuto

I molteplici elementi di incertezza che caratterizzano il quadro geostrategico non consentono di escludere che, anche nel prossimo futuro, si verifichi nuovamente la necessità di una disponibilità immediata di capacità militari idonee allo svolgimento dei compiti che, all'estero e in Italia, potranno essere assegnati, con minimo preavviso, alle Forze armate. Ne consegue che il Parlamento, se da un lato delibera la partecipazione delle Forze armate alle missioni internazionali, ha la precisa responsabilità di garantire che queste siano adeguatamente equipaggiate per fronteggiare la minaccia esistente. È ovvio che questo processo di ammodernamento deve essere lungimirante. Per progettare e costruire un moderno velivolo da combattimento servono oltre dieci anni. Non sono prodotti che possano essere acquisiti al momento del bisogno. Quindi, non abbiamo solo la responsabilità di decidere se andare o no, con le nostre Forze armate, nelle missioni per la sicurezza internazionale, abbiamo anche la responsabilità di consentire al Parlamento negli anni a venire di poter sovranamente scegliere se impegnarsi o no in un intervento di gestione della conflittualità internazionale. Perché quella scelta possa effettivamente compiersi dobbiamo essere noi, oggi, ad assicurare un processo di ammodernamento delle dotazioni militari che sia stabile e proiettato in avanti. la disponibilità della componente aerotattica delle Forze armate risulta fondamentale per il successo di qualunque strategia di difesa, sia essa di pura dissuasione nei confronti di un'aggressione piuttosto che di imposizione di misure volte a ripristinare la pace e la sicurezza nel sistema internazionale. Nel corso di tutti i più significativi conflitti degli ultimi anni la componente aerotattica ha giocato un ruolo centrale nella condotta delle operazioni, risultando talvolta capace di risolvere la fase militare dello scontro e fornendo comunque, in ogni circostanza, un contributo fondamentale alle operazioni. La componente aerotattica delle Forze armate italiane è oggi costituita dai reparti equipaggiati con i velivoli progettati addirittura negli anni Settanta e introdotti in servizio negli anni Ottanta. Parte dei velivoli acquisiti sono andati perduti nel corso degli anni, per il normale degrado operativo che caratterizza ogni equipaggiamento militare. Altri velivoli sono stati radiati, in considerazione della obsolescenza tecnica e della antieconomicità di eventuali programmi di ammodernamento. Periodici aggiornamenti sono comunque stati implementati su una parte della flotta complessiva, consentendone tutt'ora l'impiego. Per questo, in considerazione dell'approssimarsi della fine della vita operativa dei velivoli attuali, l'Italia ha selezionato il velivolo F-35 quale sistema in grado di rimpiazzare i Tornado e gli AMX dell'Aeronautica e addirittura gli AV-8B della Marina, conseguendo sia un adeguamento delle capacità operative alle esigenze correnti, sia un sensibile abbattimento dei costi. A fronte delle 254 macchine acquisite in passato, si prevede infatti di acquisire solo 90 velivoli F-35 in due sottoversioni, 60 F-35A e 30 F-35B, da assegnare alle Forze armate. Attraverso la partecipazione industriale al programma F-35, l'Italia sta acquisendo un ritorno in termini di coinvolgimento del nostro sistema tecnologico e produttivo, correlato direttamente al grado di competenza e competitività che esso è e sarà in grado di esprimere in un contesto competitivo globale. Difatti, oltre che garantire un forte coinvolgimento dell'industria nazionale nell'assemblaggio del velivolo, la FACO si presta ottimamente a divenire un centro di manutenzione e di aggiornamento dei velivoli in servizio, non solo nelle Forze armate italiane, ma anche presso gli utilizzatori europei e nella regione mediterranea. Grazie al coinvolgimento del nostro sistema industriale, sia la grande industria sia la piccola e media realtà, diffusa su tutto il territorio nazionale, l'Italia sta già ricevendo un importante ritorno, sia tecnologico sia occupazionale. Il programma F-35 è importantissimo perché, finalmente, ci consente di sostenere attività industriali di altissimo contenuto tecnologico. Se decidessimo di interrompere tale programma, ci assumeremmo quindi un'enorme responsabilità di fronte alle prossime generazioni, perché avremmo precluso tante opportunità di crescita e di lavoro altamente qualificato di un serio e partecipato confronto sui temi della politica di difesa. Dal 2002, con il dibattito sul documento dell'allora ministro della difesa, Martino, da cui scaturì il superamento della leva obbligatoria, il Parlamento non ha più avuto modo di confrontarsi adeguatamente sul tema di quale modello di difesa adottare per il Paese, mentre il nostro strumento militare è stato via via ridisegnato in molte delle sue componenti, anche in ragione del mutato scenario geopolitico e dell'insorgere della stessa crisi economica, che ha dispiegato i suoi consistenti effetti sulla finanza pubblica, soprattutto a partire dal 2008. Anche da qui nasce il difficile rapporto con l'opinione pubblica, quando si tratta di esaminare - senza pregiudizio - le questioni riguardanti il comparto militare e l'operatività del nostro sistema di difesa. Come spesso possiamo constatare, la sola dimensione degli obblighi internazionali, il nostro contributo all'assunzione di precise responsabilità della comunità internazionale per la pace e la stabilità, non è in grado di determinare quella necessaria sintonia tra gli organi istituzionali e i nostri cittadini proprio in ordine alle scelte di politica militare che comunque il Paese, e, per esso, la Difesa, è chiamato ad assumere. Vale a dire che, in assenza di un'analisi sulle finalità che intendiamo assegnare al nostro strumento militare, senza una chiara esplicitazione del disegno complessivo, dell'obiettivo verso il quale siamo diretti, ai più la politica di difesa sembra muoversi quasi solo per spinta inerziale ed essere, come pure spesso si allude, grazie a una occulta intesa tra i vertici militari e alcuni settori della politica, sorda al sentire dei richiami pacifisti o semplice garante di specifici interessi industriali. Ebbene, questa lacuna va al più presto colmata. Da questo punto di vista, l'iniziativa messa in campo dal Partito Democratico nella scorsa legislatura è stata costantemente finalizzata proprio a fare in modo che il Parlamento potesse diventare il luogo di una discussione approfondita e trasparente sul nuovo modello di difesa da realizzare anche nel quadro dello stesso processo di integrazione europea. Per tutto l'arco di quella legislatura, infatti, il Gruppo PD ha proposto l'istituzione di una apposita Commissione bicamerale con l'obiettivo di ridefinire il nuovo modello di difesa. Questa proposta non è risultata praticabile. Ciononostante, anche grazie al nostro posizionamento politico si è giunti, come è noto, all'approvazione della legge n. 244 del 2012, che tra l'altro, ricordo questo dato, prevede entro il 2024 una consistente diminuzione della forza impiegata, con il passaggio dagli attuali 190.000 a 150.000 militari. Pure quindi in assenza di una complessiva revisione del modello di difesa, il percorso segnato dalla legge n. 244 offre l'occasione per un partecipato confronto sulla stessa trasformazione del comparto. Una trasformazione già in parte in atto, considerato che la Difesa, al pari e forse più di altri settori della pubblica amministrazione, è coinvolta nei processi previsti dalla cosiddetta *spending review*. Da questo punto di vista, è utile ricordare che la spesa italiana per la difesa ha subito nel corso dell'ultimo decennio una consistente contrazione, raggiungendo la doppia cifra in termini percentuali, collocandosi ben al di sotto della media europea del comparto. A significare la portata della legge delega n. 244, basta citarne i punti principali: Da questo punto di vista, quindi, ben si comprende che le disposizioni del dicembre 2012 pongono nei fatti il tema di una possibile ricalibratura del nostro strumento militare, sia sotto il profilo delle risorse finanziarie messe a disposizione sia per quanto riguarda l'assetto tecnico-operativo. Una possibile ricalibratura da realizzare, come già detto, tenuto conto del radicale mutamento dello scenario geopolitico, così come del processo di integrazione della difesa europea, che avrà una sua importante sede di discussione nel prossimo Consiglio europeo di dicembre. Siamo in presenza, quindi, signora Presidente, di oggettive condizioni normative e politiche che possono determinare una possibile revisione dello strumento militare, senza, con questo, mettere in mora le prerogative degli organi istituzionali interessati, in particolare dell'Esecutivo e del Parlamento. Questo è l'approccio da assumere: considerare cioè il complesso delle questioni allo scopo di meglio indirizzare ogni decisione riferita alla eventuale revisione del nostro strumento militare, che può essere pienamente compiuta solo con l'eventuale ridefinizione del nostro modello di difesa. Il Parlamento resta la sede dove si dovrà assumere ogni decisione di quadro e dove sarà possibile sviluppare ogni utile e necessario approfondimento anche relativamente all'acquisizione dei sistemi d'arma, secondo e in applicazione della procedura riscritta, come è noto, dalla stessa legge n. 244 del 2012, in particolare agli articoli 2, comma 1, lettera *e*), e 4. degli F-35 è giusto, quindi, far rilevare come la messa in campo di una fase di studio, approfondimento e valutazione del progetto risulti quanto mai in linea con quanto fin qui rappresentato. A quattro anni dai pareri espressi sull'argomento dalle competenti Commissioni difesa di Camera e Senato, l'ulteriore impegno del Parlamento può pertanto rappresentare un'utile occasione per meglio supportare ogni valutazione su questo specifico programma, considerate le copiose e articolate implicazioni tecnico-operative, di natura finanziaria e di politica industriale sottese all'attuazione del progetto stesso. Insomma, un po' di sano buon riformismo e meno demagogia! *(Applausi

colleghi senatori, gli ultimi due interventi dei colleghi Gualdani e Pegorer ci hanno richiamato, con molta precisione e senza fronzoli retorici,

Da questo punto di vista, nel parlamentarismo del nostro tempo ogni legittima nostalgia dei Parlamenti nei quali si contrapponevano burro e cannoni, i Turati e i De Amicis, poi Sandro Pertini (quando invece che cannoni erano euromissili), non facilita l'acquisizione della centralità del Parlamento.

institute*", tutt'altro che filoatlantista e antipacifista. Secondo questo centro, la spesa militare in Italia

(era l'arco di tempo che prendeva in considerazione poco fa il collega Pegorer, evocando gli anni trascorsi dal rapporto dell'allora ministro della difesa Antonio Martino). Cioè quella del nostro Paese è di gran lunga la maggiore riduzione, l'unica a due cifre, riscontrata fra i Paesi occidentali. Questo serve a far restare, per quanto possibile, fuori gioco gli argomenti di tanta facile demagogia e anche di qualche volgarità. Mi consenta il senatore Marton di dirgli con molta franchezza che quella sua conclusione sul figlio del Ministro della difesa con la pistola in mano mi è sembrata non meno sguaiata parole pronunciate in un comizio da un altro collega, sulle quali è cominciata la seduta di oggi. Ma prescindiamo da tutto questo e cerchiamo, come sono stati capaci di fare i senatori Gualdani e Pegorer, di collocare queste mozioni nell'ambito di due scadenze: una è quella della difesa europea, il prossimo Consiglio europeo di dicembre 2013, e l'altra - mi rivolgo in particolare ai colleghi della sinistra, dell'oggi PD - è quella della grande sconfitta degasperiana del 1953, quando il Parlamento francese (presidente del Consiglio Mendès-France) non ebbe l'orgoglio e il coraggio sufficiente a porre la questione di fiducia sul tema della Comunità europea di difesa. De Gasperi ne morì addirittura di dolore e sono sicuro che nella sensibilità di un degasperiano di almeno tre generazioni successive, l'amico Ministro della difesa, questa è una preoccupazione costante, che lo ha portato a trovare una faticosa mediazione, tre settimane fa, alla Camera dei deputati e gli impone oggi in Senato un ulteriore passo avanti. Colleghi della sinistra, colleghi del Partito Democratico, non voglio essere sciacallo e non lo sarò mai sulle questioni interne. È evidente che c'è una componente di pacifismo, di antiamericanismo, di antioccidentalismo, chi sia sia al Governo del Paese. Però voi non potete bypassare il fatto che qui partiamo da una storia che comincia con uno dei vostri padri fondatori, quando ministro della difesa non era il liberal-liberista Antonio Martino, ma un uomo del cattolicesimo sociale, Beniamino Andreatta: entrambi avevano quelle categorie dell'occidentalismo, dell'europeismo come altra faccia dell'atlantismo e non dell'uno per giocare a *ping*-*pong* contro l'altro. da questo punto di vista il nostro Gruppo si schiera con piena adesione a favore della mozione presentata dal e sulla quale c'è anche la firma del nostro capogruppo Ferrara. Ci auguriamo che sia approvata. Ci auguriamo che essa possa onorare quella centralità del Parlamento che non onora invece quell'atteggiamento di parlamentarismo alla Trotzkij: la criticità permanente in nome dei valori della pace. è retorica di maniera e non sempre di buon gusto. Però non si sfugge, con una difficoltà rispetto alla propria storia, accelerando qualche mozione di sfiducia inopportuna prima che si sia pronunziata un'inchiesta richiesta dal Presidente del Consiglio.

senza alcun tatticismo, con gli stessi sentimenti con i quali, quando c'erano Prodi a Palazzo Chigi e D'Alema al Ministero ci siamo schierati con le mozioni in difesa dell'atlantismo aventi per oggetto la base americana di Vicenza e su tante altre. E siccome non ci piace il tatticismo, meno che mai in politica della difesa, che senso ha opporsi e dilazionare, in nome di una specie di trotzkismo parlamentare, un progetto che è

Sarebbe un argomento legittimo, anche se io non lo condividerei; ma già so le urla di sionismo, di israelismo e di quant'altro verrebbero dagli stessi colleghi

Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, la ragione per la quale sosterrò la sospensione non è legata alla considerazione che la pace si protegge con la fionda o con l'arco e le frecce. Non è mai successo nella storia, né recente, né lontana: la pace si difende con gli strumenti della diplomazia e molte volte la si è protetta, nella storia, anche con le armi.

L'Italia, con il crollo e le difficoltà della sua spesa pubblica e con il suo stato di straordinaria difficoltà, è obbligata a scegliere, non potendo fronteggiare una pluralità di impegni assunti nel tempo. Vanno quindi definite meglio le priorità intorno alle quali costruire consenso e costruire una credibilità parlamentare. Poi c'è una ragione diversa, che è invece di ordine militare. Prima ancora che dibatterla all'interno del Parlamento italiano, e oggi del Senato, essa è stata sollevata da Paesi che avevano assunto, prima di noi, impegni più forti di quanto non ne avesse assunti il Governo italiano e si lega alla domanda se si tratti ancora di un programma adeguato - quello di cui stiamo discutendo, signor Ministro e se si tratti di un programma che sia legato al futuro o sia, invece, un passo nel passato prossimo. Lo hanno richiesto e hanno fatto sì che questa domanda avesse una sua verità tre grandi questioni legate a Paesi che hanno sottoscritto con noi - anzi, hanno sottoscritto prima di noi - impegni ancora più vincolanti. Primo tema: la maggior parte dei Paesi che appartengono alla NATO - lo sappiamo già - non adotterà più questi velivoli. La seconda questione coinvolge un *partner* primario della NATO e dell'Europa, la Gran Bretagna, che taglia drasticamente questo impegno di spesa. Poi vi è una ragione oggettiva, che riguarda l'Italia, la quale ha un impegno, nell'acquisto dei velivoli di cui stiamo discutendo, non ancora formalizzato. Il senatore Di Biagio ci ha giustamente richiamati a discutere in concreto del tema. Ricordo al senatore Di Biagio - lo faccio volentieri - che i fatti che ora ho ricordato, questi tre fatti, sono fatti oggettivi che conviene tenere di fronte a noi prima di assumere ogni e qualsiasi altra decisione. Aggiungo - e confermo una posizione che so essere cara al Ministro che segue questo dibattito - che occorre muoversi nel concerto di una posizione comunitaria, e quindi nel concerto di una posizione condivisa in Europa. sosterrò la tesi del sospendere per rivedere e dell'investire in un progetto condiviso all'interno della difesa europea. L'ultima nota mi permetto invece di sottolinearla legandola a quei giuristi decisamente troppo frettolosi ed eccessivamente realisti che hanno (ma è la mia opinione) mal consigliato il Presidente della Repubblica. Lo faccio ricordando a noi e a loro che il Senato della Repubblica non è mai stato e non è (per lo meno non dal 1948 in poi) una sorta di *consilium regis*: è un organo che ha la sua autonomia,

che spetta al Parlamento definire la copertura di bilancio: spetta a noi e soltanto a noi, non ad un altro organo previsto dalla Costituzione italiana. luogo spetta al Parlamento, come si scrive nella mozione, definire il «cosa», il «come» e il «quando», come compete a tutti gli organi sovrani, dotati di potere sovrano. Se nella mia esperienza universitaria avessi sostenuto un esame rispondendo con il criterio utilizzato da quei giuristi, il mio libretto, come diceva un grande docente che ho avuto la ventura di avere, il professor Cheli, sarebbe - come sosteneva lui - volato dalla

ma cercando di ricostruire una vicenda che impegna il Parlamento italiano da tempo, da anni e che hanno evidenziato quanto questa vicenda sia nata male.

Parliamo infatti di un mezzo, care e cari colleghi, smaccatamente offensivo. Evitiamo di arrampicarci sugli specchi,

pericoloso non solo per chi lo subisce, ma anche per chi lo usa. Sono altre le priorità che anche dagli ambienti militari emergono, legate sia al sistema difesa in generale sia alla sicurezza dei nostri militari.

Anche nel campo delle spese militari questo eventuale impegno comporterà che non potranno essere assunte altre misure legate alla difesa

Non possiamo permetterci di toccare risorse essenziali che debbono - non possono: debbono - essere impegnate per fondamentali emergenze. Lasciamo perdere poi le considerazioni - quelle sì di natura ideologica - in merito a un complotto internazionale, all'antiamericanismo che albergherebbe nelle fila di una certa sinistra. State tranquilli: fosse fatto da chiunque questo mezzo sarebbe da noi stigmatizzato assolutamente allo stesso modo, seppure di più, così pure se fosse sostenuto dallo stesso o contrario schieramento politico.

è amara la considerazione che avete fatto. Non solo non convince, ma sposta tutto dal terreno del merito a quello della drammatica compravendita di voti.

presuppone l'impossibilità di praticarne altre, anche sulla carne viva del nostro Paese. Insieme ad altri parlamentari del Partito Democratico, venerdì a visitare la più importante caserma dei Vigili del fuoco di Roma e di una vasta area del nostro Paese, con sede a Capannelle.

Forse basterebbero poche centinaia di migliaia di euro, che potrebbero diventare qualche milione su scala nazionale, per far fronte ad eventuali tragedie che possono colpire il nostro Paese. Paese. Di questo parliamo. Pochi giorni fa, il mese scorso, non abbiamo dato le risposte almeno sufficienti alle emergenze terremoto dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna. Non è demagogia: è dire facciamo delle scelte o facciamone altre. Se siamo nella piena responsabilità, come da tutti è stato ricordato, contrariamente ad alcune interpretazioni

parlassimo di un futuro in cui dovrà svolgersi un dibattito. Ecco: un dibattito è un pronunciamento del Parlamento. È importante che, in una discussione come questa, possa essere incanalato o introdotto un chiaro indirizzo.

di fare questo dibattito e di prendere qualche decisione coerente in merito. Sui valori fondamentali non ci possono essere trattative, non ci può essere *realpolitik*: ha già fatto troppi danni, ha causato troppi lutti e rovine. Liberiamoci dalla schiavitù - diciamolo - della potente *lobby* degli armamenti. Ci vuole coraggio: lo sta esercitando Obama questo coraggio, non possiamo farlo mancare noi. Non ci dite che non porta voti, perché per la pace bisogna starci, senza se e senza ma e, soprattutto, senza però.

momenti così difficili per l'economia, per la gestione dell'ordinario dei bilanci pubblici, ma anche di quelli delle famiglie italiane. In un momento come questo, parlare di cifre importanti investite nella difesa indubbiamente fa sorgere tante domande: Ci sono settori a cui dare priorità, cui indirizzare queste risorse? Indubbiamente si tratta di visioni tutte legittime e tutte degne di ricevere attenzione. se non si vuole solo cavalcare demagogicamente la questione ci dobbiamo porre poche domande. Cosa è la difesa oggi? In un contesto come l'attuale, la difesa non è più vista come

addirittura dell'ONU) in cui le varie componenti delle difese di ogni singolo Stato partecipano nei limiti delle capacità e dei contributi che possono dare alle operazioni. Operazioni di quale natura? Il primo grande nemico dell'Occidente oggi è un nemico invisibile: è il terrorismo internazionale. Lo devi arginare dove si forma, si organizza, si addestra, perché quando è a casa tua non lo vedi più e subisci soltanto atti Il Mediterraneo è lo scacchiere regionale più caldo che esista in questo momento: vi è una guerra civile in Libia; Libia; conosciamo il travaglio che sta passando l'Egitto; la Siria è in pieno tumulto. Insomma, che si fa? Si può stare a guardare, sperando che tutto rimanga entro confini più o meno nazionali? C'è la necessità di avere a questo punto organizzazioni di difesa in grado di tamponare queste situazioni, che sono di pericolo interno ancorché combattute magari a decine di migliaia di chilometri.

più vetusti che esistano; abbiamo mezzi che hanno trent'anni, altri quaranta, e dovendo combattere, dovendo partecipare ad operazioni interforze, rischiamo di venire messi in un angolo perché non solo non siamo utili, ma rischieremmo quasi di divenire noi di divenire noi non più i soccorritori ma quelli da soccorrere, in quanto mezzi di una certa vetustà non danno le garanzie che dovrebbero dare. c'è la necessità di un ammodernamento dei nostri mezzi; c'è la necessità di garantire la sicurezza ai nostri militari. C'è poi la volontà politica - questa si può discutere - se voler fare parte di quella componente di Paesi che hanno un certo peso politico ed economico o se questo non interessa, e ognuno si fa gli affari propri. Questo progetto vede coinvolti i massimi Paesi industrializzati del globo: Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Gran Bretagna, oltre che Norvegia, Turchia, Olanda. Il ruolo dell'Italia,

Noi potevamo anche decidere di andare a comprare aerei da chi li produce, oppure mettere in *pool* questa importante *joint venture* di grandi forze, di Stati che hanno una tradizione di difesa militare considerevole, e in questo progetto partecipare alla realizzazione con le nostre aziende della difesa. Questa è stata la scelta, che ormai ha più di dieci anni,

(Napoli), l'Alenia di Foggia e particolarmente l'Alenia Aermacchi di Cameri. Per ora un progetto che darà 1.500 nuovi posti di lavoro, ma che arriveranno a più di 10.000 con le ricadute e il coinvolgimento di tante industrie italiane di straordinaria capacità, discussione) valore aggiunto, che investono moltissimo in ricerca, portando prestigio italiano, ma soprattutto lavoro italiano. Di questi aerei se ne realizzeranno più di 4.000. Ebbene, noi non abbiamo questa forza (a Cameri probabilmente riusciremo a sfornare circa due aerei al mese), ma in Italia si faranno le fusoliere e le ali, che sono le componenti forse più importanti di questo mezzo. Di più: a Cameri vi sarà di fatto l'assemblaggio finale l'assemblaggio finale (il FACO) di tutti questi aerei e il centro di manutenzione per tutti gli aerei che verranno venduti in Europa alle Marine e alle Noi dobbiamo cambiare tutti gli Harrier della Marina, gli AMX e i Tornado, almeno quelli che hanno passato il trentennio di vita. già all'orecchio qualcosa non suona molto bene, ma se vogliamo ricordare quanto accaduto in Libia, la partecipazione italiana è stata importantissima;

È probabile che, essendo questo un aereo di quinta generazione, difficilmente vi saranno aerei che supereranno come concezione quello di cui si sta parlando, ma è probabile che arriveremo a costruire aerei molto, molto più costosi, che non saranno neanche più pilotati da una persona, ma saranno a pilotaggio remoto. I droni esistono: per ora sono ancora piccoli e hanno funzioni limitate, ma la strada sarà questa. Dovremo essere ancora più disposti a spendere, a fare investimenti ancora maggiori, a garanzia però che non vi saranno più vite umane esposte Pertanto la domanda, se vogliamo essere corretti e onesti, deve essere questa: serve all'Italia un esercito? Prima domanda. Serve all'Italia avere un'aviazione? Seconda domanda. Se sì, dobbiamo anche essere all'altezza, sia dei tempi sia delle alleanze e di quello che ci si chiede. Altrimenti, ed è questa la scelta politica, possiamo anche decidere di fare come si fa in Svizzera. Noi riteniamo, in conclusione, che fra tutte le posizioni espresse, l'unica che può essere condivisibile è quella contenuta

Presidente, colleghi, comprensibilmente, la gravissima crisi economica nella quale si dibatte il Paese ha dato maggior vigore alle forze che chiedono una riduzione delle spese militari.

militari. Meno comprensibile è la campagna contro la produzione e l'acquisizione dei velivoli da combattimento che, in numero drasticamente ridotto, dovranno sostituire ben tre tipi di sistemi che sono in servizio da decenni e il cui mantenimento in decorose condizioni operative sta sta diventando sempre più oneroso e sempre più problematico, specie se si considera che è passato soltanto un anno dal dibattito parlamentare sugli aerei militari F-35, durante il quale il Governo Monti ha comunicato la decisione di ridurre il numero dei velivoli che l'Italia intende acquistare da 131 a 90 e il Parlamento ha respinto le richieste di sospensione e di cancellazione del programma. Una campagna difficile da comprendere, in primo luogo perché appare sotto esame uno solo dei programmi di investimento della Difesa. Coerenza vorrebbe che gli ambienti antimilitaristi e pacifisti considerassero, ed eventualmente mettessero in discussione, anche altri tipi di spesa militare. La pregiudiziale ideologica emerge chiaramente nella menzione del fatto che l'acquisizione, testo di una mozione, rischierebbe di compromettere le politiche di disarmo. Sarebbe interessante sapere quale programma di sviluppo militare sia compatibile con il disarmo. Se questo è l'obiettivo, bisognerebbe proporre lo smantellamento delle Forze armate e non la cancellazione di uno dei programmi di acquisizione. Campagna difficile da comprendere, in secondo luogo, perché l'argomento finanziario si basa sull'assunto, totalmente infondato, che ci siano oggi, da qualche parte, nelle casse delle Difesa 15 miliardi accantonati per gli F-35 che potrebbero essere dirottati verso programmi socialmente più desiderabili (come l'edilizia scolastica o gli asili nido) e che il mancato reperimento di risorse per la scuola e il territorio sia legato a una spesa eccessiva per l'acquisizione di materiali di difesa, quando invece tale spesa incide complessivamente per meno dello 0,5 sulla spesa totale annua dello Stato e ridurre ulteriormente un capitolo di spesa così esiguo non consentirebbe di migliorare la tenuta idrogeologica del territorio e, in cambio, avrebbe conseguenze disastrose sul dispositivo di difesa nazionale. Va da sé che un dibattito pubblico trasparente e informato non può che migliorare la qualità delle scelte in materia di armamenti: a condizione, però, di affrontare la questione senza i pregiudizi ideologici che dominano il dibattito in corso. Se si parte dalla convinzione che il possesso di materiali di difesa sia immorale, come è stato detto, non è possibile una valutazione oggettiva della opportunità di aderire a un programma. Il dibattito però serve, specie se considera che è in corso un attento riesame dello strumento militare nel suo complesso, finalizzato a definire le esigenze nel quadro strategico attuale e in quello ragionevolmente prevedibile, per poter disporre di quello che occorre non solo e non tanto in ambito nazionale, quanto in vista di un futuro, anche se non prossimo, processo di integrazione della difesa europea. Un riesame mirato a rimodellare le nostre Forze armate, sebbene ridotte nei numeri, in modo da avere uno strumento equilibrato in tutte le sue capacità e componenti, utilmente impiegabili a sostegno della politica estera e nazionale. Le cose da chiarire a livello politico sono parecchie, a partire dalla definizione esatta dello strumento militare del quale il Paese si deve dotare e dei suoi obiettivi, come ha riconosciuto lo stesso ministro Mauro, anche in vista del Consiglio europeo del prossimo dicembre, che per la prima volta si riunirà anche nel formato Ministri della difesa. Ciò comporta una valutazione della posizione e della forza della NATO, che oggi è erosa dalla lenta deriva statunitense. Comporta un giudizio circa la riluttanza dell'Unione europea ad organizzarsi credibilmente in termini di sicurezza e di difesa, aggravata dalla sempre più evidente tendenza britannica a defilarsi da ogni impegno comunitario. Comporta una valutazione della sicurezza delle fonti energetiche e del continuo palleggio di responsabilità tra NATO e Unione europea, il che aiuterebbe a capire che cosa ci stavano a fare due marò italiani a 20 miglia dalle coste indiane. Comporta una valutazione dei concetti su cui si impernia la cosiddetta responsabilità di proteggere. O l'abbiamo dimenticata? Dimenticarla significherebbe che noi non vogliamo la pace; vogliamo semplicemente essere lasciati in pace,

e se deve, come prescrive l'articolo 11 della Costituzione» - basterebbe leggerlo per intero - «cooperare, in condizioni di parità con gli altri Stati, per assicurare la pace e la giustizia

L'argomento che, trattandosi di un sistema prevalentemente concepito per l'attacco al suolo, sarebbe in contraddizione addirittura con il dettato costituzionale, confondendo il livello politico‑strategico con quello meramente tattico, è inconsistente solo che si consideri anche il secondo comma dell'articolo 11. Proprio gli avvenimenti della crisi libica dovrebbero farci riflettere: davvero i mezzi militari ad alta tecnologia sono inutili e non impiegabili? Siamo proprio sicuri che il contesto internazionale rimanga quello in cui l'unico utilizzo delle Forze armate appariva quello delle missioni di *peacekeeping*, senza dover ricorrere alle forme di impiego definite ad alta intensità? Siamo sicuri che questo contesto non sia destinato a cambiare e non sia già cambiato? Anche perché non possiamo illuderci che il domani sia uguale a quello che accade oggi. E in assenza di una capacità di garantire alle truppe sul terreno la copertura aerea, l'Italia si vedrebbe ridotta a fornire *boots on the ground*, le truppe sul terreno, da mettere a disposizione di altri, confidando sulla volontà altrui di sostenere e di proteggere le nostre unità. Il mondo sta cambiando vorticosamente, ma un paio di cose le conosciamo. Sappiamo ad esempio che esempio che ci sono alcune costanti storiche destinate a pesare per il nostro Paese in qualunque contesto interno e internazionale. La prima ha a che fare con la vulnerabilità e l'insicurezza, a causa del debole assestamento e della continua instabilità instabilità di due versanti obbligati della politica estera italiana: la penisola balcanica e la sponda Sud del Mediterraneo. L'altra costante, che ha costituito e per molti versi continua a costituire una risposta a questa prima condizione, è l'ancoraggio alle alleanze bilaterali o a sistemi di alleanza con attori più forti, in grado di colmare il *deficit* di sicurezza, internazionale e qualche volta anche interno. Grazie a questa politica di alleanze, l'Italia ha raggiunto importanti obiettivi, a cominciare dalla stessa unità nazionale. Questa politica ha naturalmente anche dei costi. Ora le cose stanno cambiando. La crisi economica, la distribuzione del potere su scala globale, il lento spostamento del baricentro politico, strategico ed economico del sistema internazionale verso l'Asia,

l'indebolimento dell'opzione multilateralista, sulla quale l'Italia ha fondato la propria politica estera all'indomani del trauma della guerra, proprio oggi che i problemi che gravano sulla sicurezza sarebbero tali da richiedere risposte concertate, risposte multilaterali. Ciò vale per la crisi del debito come per la guerra civile siriana. Su questo converrebbe riflettere; visto il posto che l'Italia occupa nella gerarchia del potere, non ci sono alternative credibili. Anche per questo bisognerebbe cercare di limitare i danni di una campagna di disinformazione che è stata condotta in questi termini, favorendo invece una riflessione che abbia consapevolezza delle implicazioni e dei relativi costi. I veicoli per l'attacco al suolo, di cui si è parlato, sono già serviti al nostro Paese in maniera limitata per colpire obiettivi militari durante l'intervento in Kuwait, durante l'intervento in Kuwait, in Kosovo, in Iraq, in Afghanistan ed in Libia, a protezione della popolazione civile, delle loro nuove forze di sicurezza e dei nostri uomini. Potrebbero un domani servire a proteggere anche la nostra comunità, e un Paese che vuole avere una minima capacità di difesa non può rinunciarvi. Più in generale, sembra esservi un'eccessiva confusione di ruoli; spetta ai tecnici indicare la strumentazione loro necessaria. Non si possono indicare ai Vigili del fuoco i mezzi di cui devono dotarsi per spegnere gli incendi e non lo si dovrebbe fare nemmeno con i militari italiani.

il dibattito sugli F-35 permette di rimarcare ulteriormente lo spartiacque tra chi pensa alla pace come un obiettivo da costruire con tutte le forze e in verità e chi, invece, si richiama a parole alla pace per costruire comunque una cultura di guerra. Ho un ricordo ancora fresco delle parole dell'attuale ministro della difesa Mauro, mi sembra sia di formazione cattolica, secondo cui per amare la pace bisogna armare la pace. Ricordo che proprio 50 anni fa il pontefice Giovanni XXIII dava alle stampe un'enciclica che da questo punto di vista ha illuminato, prima che le menti, i cuori di mezzo mondo. Mi riferisco papa Roncalli sosteneva che il vero promotore di pace non può che essere l'uomo di giustizia, per cui piuttosto che armare la pace, bisognerebbe quindi costruirla facendo giustizia. Questi discorsi sono certamente impegnativi per chi reputa invece che, in un momento di disperata crisi sociale ed economica, sia preferibile fare spese enormi, abnormi per l'acquisto di cacciabombardieri che, a giudizio di chi li dovrà anche pilotare, non sono affidabili. Si tratta inoltre di velivoli prevalentemente d'attacco,

contrastare le politiche di guerra significa investire in sviluppo, che però sia rispettoso della dignità e delle culture degli altri popoli e degli altri Paesi. Rammento a me stesso, e questo è un ricordo che propongo a tutte le parti del Parlamento, che noi in qualche occasione passata ci siamo fatti coinvolgere in guerre preventive. sul concetto di guerra preventiva bisognerebbe ragionare. Ricordo ancora che in campagna elettorale tanti - e molti sono presenti in quest'Aula - si sono espressi contro l'acquisto degli F-35 e contro la realizzazione di un programma che di pacifico non ha assolutamente nulla. Ricordo infine, perché mi piace essere molto semplice nelle mie considerazioni, che chi adesso si accompagna a certe *lobby,* che vorrebbero si procedesse alla realizzazione e all'acquisto di questi strumenti di guerra, magari qualche anno fa, alla fine degli anni Novanta, canticchiava una canzoncina, «Il mio nome è mai più», che presso tanti giovani voleva significare il rifiuto di una cultura di guerra. Una cultura di guerra che tuttavia ancora oggi ci ostiniamo a praticare, perché poi, alla fine, quando c'è da incassare e da monetizzare,

continua a far soldi senza che gli vengano tassati, senza che possano essere oggetto di un intervento precipuo. Sappiamo infatti che c'è un commercio internazionale di armi contro cui a parole ci battiamo, ma che di fatto continua a prosperare. Vi ringrazio, sono convinto della vostra attenzione.

dell'organico da 190.000 a 150.000 unità, come è stato ricordato: parliamo di donne e di uomini, di servitori dello Stato che non potranno più assolvere questo compito, parliamo

Ebbene, quando nel 1998 (il ministro della difesa era Scognamiglio Pasini), fu avviato questo percorso, vi furono una riflessione seria e un'indagine conoscitiva per capire la validità e la valenza del progetto. Credo che quando parliamo di dimensioni globali ed internazionali, l'Italia - quella che ancora accetta le sfide - non si debba e non si possa sottrarre: non possiamo continuare a fare un passetto avanti e due passetti indietro.

Parlai con il ministro Agnelli, quando Sarajevo era un macello all'aria aperta, dove uomini, donne e bambini erano sotto il tiro dei cecchini. Persero la vita a centinaia. Mi vengano in mente Srebrenica e la pulizia etnica. Cosa chiese il Papa, allora, all'Occidente? Di intervenire militarmente

diversi Governi italiani che sono accorsi alla richiesta di pace, di democrazia e di rispetto per le donne. Ricordiamo infatti che in Afghanistan le donne vengono uccise se vogliono mandare i bambini e le bambine

di ragioni. Politicamente hanno assolutamente ragione il Ministro e il Parlamento: l'Italia non può non avere una forza armata collegata alle Nazioni Unite e all'Europa, per poter essere fattore di pace e di stabilità anche nel Mediterraneo.

da 30 anni a questa parte. La tecnologia spaziale e quella militare ci hanno fornito l'informatica, i telefonini, il tempo reale; ci hanno fornito quel progresso scientifico su cui possiamo ancora essere concorrenziali con tre quarti del mondo. Se abbandoniamo anche la ricerca scientifica e gli investimenti in quel settore, cosa rimane all'Italia occupazione ai giovani ed evitare la disperazione agli adulti? Le lavorazioni che là fanno spendendo un centesimo di quello che spendiamo noi? Pertanto, anche da questo punto di vista, dire di no alla ricerca avanzata è un suicidio per il Paese. Sono quindi solidale con il Ministro e voterò con convinzione una mozione che giustamente chiede che si prenda qualche mese di tempo per approfondire la questione e fare la scelta migliore possibile per il nostro Paese.

ed è il dubbio che ci attraversa tutti rispetto a un passaggio così delicato come è quello di un investimento importante in un sistema d'arma. Il dubbio ha vari livelli e vari strati. C'è innanzitutto un dubbio tecnico: è lo strumento migliore possibile? C'è un rapporto congruo tra il costo, che è indubbiamente rilevante (stiamo parlando di 500 milioni l'anno per diversi anni), e la sua resa dal punto di vista tecnico e tecnologico? C'è il dubbio sull'utilità di questo strumento d'arma in un contesto di tipo strategico. C'è anche il dubbio che attraversa tutti gli schieramenti di questo Senato, e certamente il Partito Democratico, sulla congruità morale di un investimento di questo genere rispetto all'articolo 11 della Costituzione, e ancor più rispetto al momento che il Paese attraversa. Il Parlamento ha il diritto di esprimere questi dubbi a nome del Paese, perché questi dubbi attraversano il Paese, e ha il dovere di chiedere al Governo una verifica seria e approfondita di questo programma d'arma. Naturalmente deve esercitare questo diritto-dovere sapendo che nemmeno il potere del Parlamento è assoluto: la nostra Costituzione non prevede poteri assoluti di nessuno, nemmeno del Parlamento. E infatti il Parlamento stesso nella scorsa legislatura ha varato la legge n. 244 del 2012 che proceduralizza questa operazione, cioè stabilisce come devono essere fatte queste verifiche, perché naturalmente anche il Parlamento deve esercitare la sua funzione con responsabilità, dato che quando si parla di investimenti pluriennali non si può cambiare non si può cambiare idea per motivi futili ad ogni stormir di fronda. Se si deve cambiare idea, lo si deve fare attraverso una procedura molto seria; quando si fanno investimenti importanti, diciamo pure molto impegnativi, con altri Paesi, a livello internazionale, c'è in gioco anche la credibilità del nostro Paese e quindi è necessario che le verifiche che le verifiche vengano fatte salvando quest'altro valore che comunque è in gioco. Su questo siamo uniti, cari colleghi, e lo vorrei dire in modo particolare - mi dispiace che non ci sia il collega Casson - ai colleghi del Partito Democratico che hanno deciso e stanno decidendo di mantenere una loro mozione, che loro dicono essere in realtà molto simile a quella della maggioranza, il che rende non del tutto comprensibile la loro scelta. C'è un punto, invece, che ci differenzia, che - non me ne vogliano i colleghi - a me suona di propaganda, è quando il dubbio cede lo spazio alla propaganda: perché mentre nel dubbio siamo uniti, vorrei che evitassimo la caduta del dubbio nella propaganda. È la propaganda che lascia intendere che ci sarebbero miliardi di euro disponibili per asili, scuole, ospedali, assetto del territorio se solo si accettasse di tagliare un po' il grasso bilancio della difesa italiana. Le cose, cari colleghi, non stanno così, e lo sappiamo tutti. Basta leggere non i documenti ufficiali della difesa ma - è stato già citato - il documento di Archivio Disarmo: per arrivare a un punto percentuale di PIL, l'Archivio Disarmo mette dentro i costi della Difesa anche le pensioni del personale militare. E io non voglio discutere sulla correttezza, mi va bene: basta che sappiamo di cosa stiamo parlando. Quindi, le cose non stanno così. Sono anni che il bilancio della Difesa viene tagliato in proporzione più di ogni altro comparto della spesa pubblica. Oggi l'Italia spende per la difesa lo 0,85 per cento del PIL, pari a circa 13 miliardi di euro l'anno, su 800 miliardi di spesa pubblica complessiva. Nessun altro Paese occidentale spende così poco. E io dico che questo è un valore, è un fatto positivo: vuol dire che l'Italia ha fatto una scelta certamente non di riarmo. Ma è di questo che dobbiamo parlare, non di una inesistente corsa agli armamenti. Non è tutto. Questi 13 miliardi per il 70 per cento sono stipendi dei militari e per il 10 per cento (troppo poco) spese di esercizio, mentre solo il 20 per cento è impiegato per gli investimenti, ossia per l'acquisto di sistemi d'arma. Siamo al di sotto del livello minimo di mantenimento in efficienza del nostro apparato militare. Anche le macchine militari, come tutte le macchine, si tratti di carri, navi o aerei, invecchiano fino ad andare fuori uso. È quello che sta succedendo a 250 aerei militari che dovrebbero essere sostituiti nell'arco dei prossimi 15 anni da 90 F-35 (90 al posto di 250), con un investimento di circa 500 milioni l'anno, altrimenti resteremmo praticamente senza Aeronautica militare. Ho sentito dire che non si dovrebbero costruire nemmeno le fregate; quindi, resteremmo anche senza Marina

nel senso della «*Pacem in terris*» perché il Mediterraneo diventi un lago di pace, e tutta la nostra politica estera è impegnata in quella direzione. Guai se non lo fosse. Ma oggi il Mediterraneo è l'area più instabile e pericolosa del mondo, questa è la realtà con la quale ci dobbiamo confrontare, ed è probabile che resti così a lungo. In prospettiva sarà anche necessario e giusto che la difesa diventi una materia di competenza europea. Lasciate ricordare ad un senatore che si ritiene degasperiano per ispirazione l''importanza del Consiglio europeo di difesa che De Gasperi non riuscì a varare. Quel sogno è ancora il nostro sogno, ma ci vorranno anni per realizzarlo, forse decenni, e in ogni caso la nostra bolletta per il costo della difesa difficilmente potrà ridursi, essendo oggi la più bassa d'Europa. In conclusione, va bene sospendere, approfondire, verificare, cercare di ridurre e di rimodulare, ma non vendiamo illusioni a buon mercato, colleghi e amici di quest'Aula. Non facciamo questo errore. Una contenuta e ponderata politica di investimenti nel settore della difesa è a tutt'oggi indispensabile. Negare questo dato della realtà non è buona politica: è cattiva politica. Ci permettiamo di dirlo sommessamente, ma anche con fermezza, la stessa con la quale voteremo a favore della mozione

distruggendo interi raccolti di pomodoro, mais, erba medica, anguria, melone e vigneti, che sono stati compromessi probabilmente anche per la prossima stagione. Sono più di 200 le aziende colpite. Stiamo parlando di un territorio e di una provincia che già hanno

che ha colpito l'Appennino di quel territorio ed un secondo sisma nell'Appennino tosco-emiliano. Ora, infine, si è verificato un evento climatico che in 15 minuti ha distrutto intere coltivazioni. Chiedo che quest'Aula dedichi

anch'io volevo riallacciarmi a questo argomento, perché sono stati colpiti non solo i Comuni della bassa reggiana, ma anche tutta la zona del cremonese, quindi il casalasco e il viadanese. Anche lì ci sono state grandinate tremende: 10 centimetri di grandine e 60 millimetri di acqua in due ore. La Regione Lombardia, tramite il suo assessore Fava, ha già annunciato che chiederà lo stato di calamità,

Signora Presidente, nei giorni scorsi il Governo ha varato un decreto legislativo molto importante, quello sulla filiazione, che riconosce parità di diritti tra i bambini nati all'interno del matrimonio e quelli finora considerati

un percorso di ammodernamento, come dicevo, i bambini di serie A e di serie B in questo Paese esistono ancora. Esistono, perché esistono tanti bambini con aggettivi - il presidente Letta, fra l'altro, ha detto che non con aggettivi - come "straniero, "extracomunitario, "di seconda generazione"; bambini che non hanno i diritti dei loro compagni di classe e dei loro coetanei, perché mancano del diritto fondamentale della cittadinanza italiana. poi esistono ancora tanti bambini che non sono uguali agli altri proprio rispetto al tema in questione, cioè quello del riconoscimento del legame genitoriale in maniera uguale a quello degli altri bambini. Sono i figli che nascono e crescono in famiglie con genitori dello stesso sesso, che ad oggi non vedono riconosciuta nessuna forma di legame giuridico con il genitore non biologico. Rimane ancora sempre forte come unico legame quello del sangue, sia per quanto riguarda il rapporto con la propria terra, sia per quanto riguarda il rapporto con i propri genitori. Voglio sperare che il decreto legislativo varato dal far maturare più in generale la consapevolezza che, al di là di quel legame profondo e ancestrale che è il legame di sangue con il proprio popolo, la propria famiglia e la propria comunità, oggi esistono anche legami diversi e che le leggi dello Stato possono andare oltre le leggi

a nostro parere importante e grave. Due giorni fa si è verificato l'ennesimo crollo a Pompei, sito di importanza mondiale e patrimonio dell'UNESCO. sito talmente importante che ogni anno incassa circa 20 milioni di euro in biglietti (sono veramente tantissimi) e talmente prioritario che il Ministero lo ha lasciato nelle mani delle Soprintendenze, che continuano a non fare nulla da anni. Un disastro culturale figlio di una mentalità ottusa che ritiene le aree culturali archeologiche come siti da non promuovere. Quindi il *marketing*, purtroppo, non esiste. Sono passati mesi dal primo crollo, il famoso crollo che costò il Ministero al collega Bondi: il Partito Democratico indicò l'allora Ministro come unico responsabile, con una mozione di sfiducia a mio e nostro parere indegna. Da allora nulla è cambiato e l'attuale Ministro, come i suoi predecessori, ad oggi nulla ha fatto per cambiare rotta: non ci sono progetti seri, né progetti seri realizzabili.